della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***

Egli ci dice, giustamente, che è molto bello, ma questa è la stessa dinamica che sta succedendo negli *slogan*, che si limitano appunto a guardare una sola parte del provvedimento. Sì, è molto bella questa parte, peccato però che ci sia tutta una seconda parte che continua a essere taciuta. E quello che è più grave è che viene taciuta proprio ai cittadini, che stanno continuando a subire un processo evidente di manipolazione. Perché non dite la verità? Perché non dite cosa sarà questo nuovo *Premier*? Questo nuovo *Premier* sarà una persona che avrà il potere di sciogliere il Parlamento come e quando vuole il Presidente della Repubblica non potrà proferire parola e non avrà più un ruolo di garanzia, ma dovrà soltanto ratificare la scelta di questo *Premier* assoluto. Il Parlamento non sarà più libero di esprimere un voto di sfiducia. Se un parlamentare vuole votare la sfiducia, dev'essere libero di votare senza avere conseguenze, altrimenti diventa un voto condizionato potrebbe diventare una scelta conservativa. Non sarà una scelta libera, ma un tenere in piedi un Governo che il Parlamento non vuole più, perché per sfiduciarlo bisognerà tornare tutti al voto. Non si torna al voto soltanto per scegliere il nuovo *Premier*, perché lo avete collegato. Quindi, se il *Premier* viene sfiduciato, si deve tornare al voto anche per la Camera e per il Senato. il Senato. È molto bella la prima parte, ma queste cose non sono state dette. Allo stesso modo, non viene detto che nel provvedimento viene inserita in Costituzione una stortura democratica, ossia costituzionalizzate un premio di maggioranza che va a minare la rappresentatività. Ora, posso capire che le esigenze contingenti conducano a una legge elettorale che introduce un correttivo forzato e fa sì che ci possa essere un Governo di minoranza. Ma com'è possibile pensare che questo diventi addirittura un principio costituzionale? Oltretutto scritto male, perché non avete nemmeno inserito come e quando va concesso questo premio di maggioranza e non avete detto in quali limiti va concesso. State scrivendo un premio di maggioranza che è peggiore di quello che avevano previsto nella legge Acerbo, che ha consentito di avere la maggioranza in Parlamento a Mussolini. Questo perché non avete messo la soglia minima. Cosa si farà? Bisognerà correggere quello che avete fatto con una legge elettorale? Come possiamo fidarci, viste le premesse e visto che comunque vi ostinate a continuare ad affermare che si tratta di una bellissima riforma, perché si dà finalmente la possibilità ai cittadini di scegliere? Non è vero, state dicendo ai cittadini di nominare un *Premier* con poteri assoluti, state marginalizzando il Parlamento e attaccando

una riforma che continuiamo a giudicare sbagliata e pericolosa, perché interviene sulle basi della nostra democrazia rappresentativa e sul principio della separazione tra i poteri sancito dalla Costituzione. E per cosa? Per quale ragione volete piegare il buon senso e le istituzioni? Per quale ragione volete ridurre a ben poca cosa il ruolo del Parlamento? Per quale ragione volete scardinare la nostra Costituzione? Lo fate per bramosia e sete di potere e per assoggettare il nostro sistema ad una parte politica. In questo articolo si stravolge la forma di repubblica parlamentare e si introduce un ibrido che fa perno sul Presidente del Consiglio. A ben poco servono i maldestri tentativi di chi dice che questo non è un abito su misura; è un abito su misura,

che neghi l'evidenza e cioè che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio contraddice i tratti fondamentali e il senso stesso della forma di governo parlamentare. Sappiamo che Fratelli d'Italia soffre particolarmente il richiamo alla Costituzione e che sta facendo di tutto per destrutturare più o meno surrettiziamente l'impianto della nostra Carta costituzionale, nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione. Lo dimostra il fatto che si sta continuando ad evitare il confronto tra le opposizioni senza alcuna ricerca di punti condivisi. Avete scelto lo scontro muscolare, procedete a strappi. Peraltro, signora Ministra, senza

Presidente, credo che dovrebbe essere suo compito quello di garantire in primo luogo il rispetto tra le parti... *(Applausi)*. PRESIDENTE. Lo sto facendo, ma non posso sapere con chi è al telefono il Ministro e onestamente, siccome sono qui, non avevo neanche visto che fosse al telefono se lei non mi avesse avvisato. Vada avanti. Come stavo dicendo, avete scelto lo scontro muscolare. La riforma della giustizia, l'autonomia differenziata e il premierato, che cancella il principio della separazione dei poteri e colpisce il ruolo del Presidente della Repubblica, non sono una partita di poker, poker, né una vicenda che può essere giocata come un gioco d'azzardo e con tanta disinvoltura, quella stessa disinvoltura che abbiamo visto in campagna elettorale e che forse non era solamente provocata da qualche *boutade* elettorale o da un colpo di calore. Penso alla disinvoltura che ha portato a tentare di logorare il Presidente della Repubblica e di portarlo nell'agone politico, come abbiamo visto dalle battute fatte anche da alcuni esponenti di quest'Assemblea. Non sono venute risposte chiare e ferme da chi avrebbe dovuto darle, a cominciare dalla signora Ministra. Noi vogliamo ancora una volta ribadire questo nostro principio, ma oggi vogliamo fare una domanda alla signora Ministra. Stiamo discutendo dell'articolo 5, ma è possibile che lei non prenda la parola relativamente a questi temi? È possibile che non si dica nulla sul sistema della legge elettorale? È possibile che su questo non si possa avere una parola da parte del Governo? penso che la risposta a questa domanda retorica sia scontata: non volete darla questa risposta, perché non siete d'accordo nemmeno tra di voi e volete cercare di nascondere la verità il più a lungo possibile. alla conclusione, per noi queste riforme non possono essere accettate così, perché sono irrazionali, figlie di una malcelata bramosia di potere, come ho detto prima; per noi, invece, le istituzioni sono sacre, sono il principio di rappresentatività, perché lì risiedono la democrazia e la partecipazione pubblica dei cittadini; per questo devono essere accessibili, contendibili e bilanciate su una base netta di distinzione dei poteri, senza senza l'invasività di una sola figura accentratrice. Di fronte a tutto questo, ribadiamo l'invito di fondo a criticare a criticare questa proposta, dicendo ancora una volta: fermatevi.

e molto giusta. Ieri sera c'è stato l'ennesimo canguro: sono dovuto andare via un'ora prima della fine dei lavori per un impegno personale e stamattina al mio ritorno ho scoperto che stiamo 200 pagine più avanti rispetto a dove eravamo arrivati, un altro canguro, com'era già successo nel corso dei giorni precedenti. Abbiamo chiesto invano in queste ore, ma anche negli scorsi giorni, di spiegarci in anticipo quale sarebbe stato l'effetto del canguro sugli emendamenti, ma non avete voluto farlo,

Martella. Io lo trovo davvero incredibile, ma mi rivolgo anche ai miei colleghi, non so come si possa accettare tutto questo: stiamo praticamente concludendo la discussione sull'articolo 5, quindi sul cuore di questo sul cuore di questo provvedimento, e lo stiamo facendo senza che nessuno, da parte del Governo e della maggioranza, dica al Paese e non semplicemente alle forze di opposizione come si come si intende che debba essere eletto questo futuro Presidente del Consiglio e come si intende che debba essere eletto il Parlamento. Stiamo concludendo l'*iter* della riforma costituzionale in prima lettura al Senato, fra pochi minuti avremo finito, si spegnerete i microfoni e ci toglierete la voce, perché i tempi sono contingentati, senza sapere questo punto essenziale. Possiamo sapere come si elegge il Presidente del Consiglio? Qualcuno ce lo può dire? C'è la possibilità concreta, come pensiamo noi, che il futuro Presidente del Consiglio, eletto con il premierato, venga eletto con la minoranza dei voti di questo Paese? Potrà succedere? È un'ipotesi in campo oppure questo scenario non esiste? Io penso che su questo, signora Ministro, occorrano parole di verità definitive: non lo dovete semplicemente alle forze di opposizione, ma a un obbligo di trasparenza nei confronti del Paese. *(Applausi)*. Non ve la potete cavare dicendo che alla fine della prima lettura ci direte, come se fosse la gentile concessione del sovrano, quale sarà la legge elettorale. Qui non c'è il sovrano e qui non c'è nessuna gentile concessione. Qui c'è la democrazia e questa Camera merita il rispetto *(Applausi)* e di conoscere perlomeno questo punto di fondo: come si elegge il futuro Presidente del Consiglio? Consiglio? Basterà che prenda la minoranza dei voti? Quanto sarà grande questo premio di maggioranza? Posso dire a quest'Assemblea che riteniamo decisive queste domande e che pensiamo che sarebbe clamoroso se l'Italia fosse l'unico Paese al mondo in cui si può diventare Presidente del Consiglio anche prendendo la netta minoranza dei voti? Penso che su questo ci dobbiate dare una risposta definitiva, non semplicemente a me, non semplicemente alle forze di opposizione, ma - lo ripeto - al Paese. Avete un obbligo nei confronti del Paese: per favore, prendete la parola e prima che ci togliate la voce, almeno rispondete a questa domanda.

l'attenzione prestata dal Governo a questo provvedimento e in particolare dalla ministra Alberti Casellati: in realtà, si sta mettendo in atto una versione 2.0 di quanto auspicava il

i rappresentanti del popolo - ricordiamolo ancora una volta, colleghe e colleghi, anche se a voi sembra essere andato in spregio il ruolo di questo Parlamento: siamo i rappresentanti del popolo

testo, hanno avvisato della pericolosità, della sgrammaticatura di questa proposta di revisione costituzionale e dell'impossibilità che essa possa combaciare con lo spirito della Costituzione repubblicana attualmente vigente. attualmente vigente. Avevo annunciato che avrei fatto una mia battaglia per difendere il buon nome dei costituzionalisti che sono stati chiamati in audizione e che vengono a volte

Fulco Lanchester, dice che ci sono almeno sette questioni per cui questo disegno di legge a suo avviso non è adeguato ed è pericoloso: perché è scritto male sia nella forma, sia nella sostanza, rivelatrice di cattivo *drafting,* che non deriva da responsabilità dei consulenti esterni, ma dalla contrattazione in infra-coalizione; perché confligge con gli *standard* del costituzionalismo democratico; perché distrugge la collaborazione elastica tra gli organi costituzionali di indirizzo attivo; perché istituisce sostanzialmente un obbligo di mandato per i parlamentari, in palese violazione dell'articolo 67. Insomma, a me inquieta il silenzio e citando in maniera inopportuna il Poeta, direi "divina indifferenza" dei rappresentanti del Governo qui in Aula, in particolare

che quanto è successo in Francia pochi giorni fa dimostra la bontà di questa revisione costituzionale,

di Stato che c'è oggi in Francia - con la possibilità per il presidente Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale - sarebbe la conferma della bontà di questo abominio di modifica costituzionale che voi avete proposto, mentre sapete benissimo che non c'entra nulla. È una cosa completamente diversa, è un *unicum* in tutto il mondo. Io vorrei davvero sapere se la signora Ministra si vergogna di ciò che la propria maggioranza afferma, sapendo che sta dicendo una falsità costituzionale. È inaccettabile questo silenzio e il lasciar passare dei messaggi del genere, delle dichiarazioni del genere, senza riprendere la propria maggioranza e dire: attenzione, senatore De Priamo, non è proprio così. Lo *status* di Macron non è minimamente equiparabile a quello del *Premier* eletto che noi vogliamo istituire. I due istituti non c'entrano assolutamente nulla È davvero mortificante il silenzio del Governo di fronte a queste palesi falsità, interpretazioni forse dovute a ignoranza, che vengono fatte dalla propria maggioranza. abbia un po' di rispetto per quest'Aula. Restituisca, perlomeno, la correttezza testuale di quanto è scritto in questa modifica costituzionale.

Il Gruppo che rappresento ha esaurito i tempi, gli altri Gruppi stanno intervenendo, siamo anche su un articolo che è il cuore di tutta questa vicenda, ma la Presidenza ancora non ci ha detto nulla rispetto al fatto se, bontà sua, intenda consentire che questo dibattito possa avvenire nella polifonia.

codificata e cristallizzata per la prima volta, nella nostra Carta costituzionale, una regola elettorale; tale regola viene codificata attraverso un processo di attribuzione di Come abbiamo visto anche nelle scorse letture, siamo un Paese piuttosto singolare. Signora Presidente e signori del Governo, che vedo impegnati in altre conversazioni, noi siamo un Paese che, quando si vota con un sistema maggioritario,

rimpiange il sistema maggioritario ed attiva delle letture di natura maggioritaria. Questo è quello che è accaduto. All'interno di questa particolare compressione sembra che non si colga un punto fondamentale, cioè che i processi politici non possono e non devono essere surrogati dalla geometria istituzionale.

Io comprendo lo sforzo della Presidenza. Comprendo meno l'idiosincrasia che sento da una parte dell'Aula al confronto, alla chiusura e allo spegnimento del pensiero, perché questa sarà, in questo momento in cui vi sentite i padroni, la strada con la quale imboccherete il vostro declino.

la Costituzione che abbiamo in vigore non fa nessun riferimento alla legge elettorale, per una ragione molto semplice: ci sono tutta una serie di pesi e contrappesi che di fatto rendono irrilevante il sistema,

una delega in bianco. Contrariamente a quello che ha detto il collega Martella, io non sono interessato, ministra Alberti Casellati, a quello che lei pensa relativamente a come verrà eletto il Presidente del Consiglio. Sa perché? Perché è irrilevante, quanto una maggioranza successiva la potrà cambiare. Noi stiamo dando praticamente una cambiale in bianco a qualsiasi maggioranza. Ciò significa che è irrilevante quello che voi state facendo, perché la prossima maggioranza la potrà cambiare

legge. Stiamo mettendo nella Carta costituzionale una delega a una qualsiasi maggioranza che potrà cambiare le regole del gioco. È questa, a mio avviso, la cosa più grave che stiamo facendo in questo momento.

però di grave c'è anche un'altra cosa: l'ipocrisia che state utilizzando nell'inserire nell'articolo 5 il rispetto del principio della rappresentatività. Ditemi, colleghi, come fate a parlare di rispetto del principio di rappresentatività quando state costituzionalizzando il Governo di minoranza? Questo Questo nuovo *Premier*, che avrà poteri assoluti, sarà il frutto di una coalizione, quindi con programmi diversi che troveranno in qualche maniera il modo di coesistere, e di un premio di maggioranza. Voi state costituzionalizzando esattamente l'opposto di quella parola che avete inserito nell'articolo 5; allora cancellatela. Perché parlate di principio di rappresentatività? La cosa più grave è che lo state facendo in un momento storico in cui c'è una bassissima affluenza alle urne. Rendetevi conto di quanto potere state dando a una sola persona, che sarà la rappresentanza di una sola forza politica, appoggiata da altre forze di coalizione, e che riceverà un premio di maggioranza. Sarà quindi sicuramente un Governo di minoranza. Voi state sostituendo lo Stato di diritto, il bilanciamento dei poteri, la democrazia, la proposta di un ritorno primordiale all'idea di una figura paterna, come se gli italiani avessero bisogno di un padre che li rassicura, che li protegge, che fuga le loro paure, che risolve in maniera semplicistica le cose. Trattate così gli italiani? Davvero pensate che siano un popolo di minorenni? Voi state approfittando di quella fetta della popolazione che mostra fragilità. alimentate le paure, invece che sottrarli ad esse. Approfittate di una fragilità che li conduce a preferire alla loro libertà uno stato di sudditanza e il bisogno di dipendere da una figura paterna,

Per introdurre un sistema di autoritarismo che è l'antitesi esatta della democrazia. La democrazia si compie infatti attraverso il dialogo democratico. Non pensate che possa esserci un dialogo democratico all'interno di un Governo dove si faranno anche le leggi

è l'attenzione che diamo a chi sta puntando sui fatti. Cari colleghi, non ci lamentiamo se poi l'astensionismo vince, perché qui non si ascolta. Ripeto: non ascoltiamo i nostri colleghi in quest'Aula.

come se fosse il Presidente del Consiglio che scioglie le Camere, ma è il Presidente della Repubblica francese! *(Applausi)*. Ma di cosa state parlando? Voi confondete gli elettori, che sono stufi di essere presi in giro. Questo vedo sui territori, perché si dice tutto e il contrario di tutto. Quando faccio i miei interventi nei convegni parlo ormai con le vostre leggi in mano, perché altrimenti non c'è modo di venirne a capo.

a menadito. Essere descritti come parlamentari che fanno errori di *drafting* volontario è gravissimo. *(Applausi)*. Non vi rendete conto di cosa state facendo.

ma avete toccato tantissimi articoli della Costituzione impunemente, modificando tutto senza dare alcuna certezza. vogliono una certezza, non hanno certo bisogno dell'uomo solo al potere (che è quello che state cercando di fare), perché è inutile nascondere che, qualora dovesse cadere il Presidente del Consiglio, si porterebbe dietro tutto il Parlamento, un Parlamento schiavo dell'uomo solo al potere. Noi invece siamo in democrazia e vogliamo difenderla, ora e sempre.

Presidente, senatori e senatrici, come è stato detto in questo lungo dibattito, siamo nel fulcro della riforma. Non mi vorrei soffermare tanto sulla questione dibattuta dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio e del meccanismo di trascinamento dei parlamentari eletti, quanto piuttosto sul richiamo alla legge elettorale. Nel passato noi abbiamo Nel passato noi abbiamo condizionato l'approvazione da parte del Parlamento delle riforme costituzionali alla definizione delle leggi elettorali e questo non è un caso:

affrontare successivamente la legge elettorale, ma perché la legge elettorale si interseca con la riforma costituzionale, e quindi con il modello che viene scelto,

cambia ulteriormente l'assetto istituzionale del nostro Paese. Non si ha soltanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma di fatto si realizza il modello all'inglese o all'americana (tra l'altro modelli in crisi) con due partiti. la decisione sulle soglie minime rappresenta un elemento di base per quanto riguarda la definizione di una rappresentatività e della capacità di inserire le le minoranze o i partiti meno forti dal punto di vista elettorale all'interno del Parlamento. La legge elettorale, connessa alla riforma costituzionale, sia per l'indicazione del premio di maggioranza, sia per quanto riguarda le soglie, determina in modo esiziale la partecipazione attiva della popolazione

Questi aspetti non sono secondari, perché, se già da un lato abbiamo individuato molto chiaramente il primo *vulnus* di questa riforma, cioè la mancanza dei contrappesi che sono previsti in tutti i sistemi in cui vengono concentrate funzioni e poteri in mano al Presidente

verrebbero articolati con meccanismi di approvazione diversi dalle riforme costituzionali nelle leggi elettorali, che andrebbero - a colpi di maggioranza - a definire in modo netto un cambiamento totale del nostro assetto costituzionale, verso il quale ci stiamo dirigendo al buio. Noi non sappiamo dove approda questa norma e quali sono le intenzioni della maggioranza rispetto all'approdo finale, che è complesso, ma che determinerà in modo fondamentale il futuro della Repubblica.

civile, anche la democrazia nel nostro Paese, perché ha mantenuto distinto il potere esecutivo dal potere legislativo. Ora

il Presidente del Consiglio va eletto in modo distinto dalle elezioni di Camera e Senato, perché il problema è che non il

davvero troppo pesante. Io penso che i cittadini la rispediranno al mittente, come hanno fatto in altre occasioni, però vorrei suggerirvi di provare ad

problema dell'elezione diretta, quella che dà la certezza e la stabilità del Governo. La stabilità c'è se c'è una maggioranza: io, ad esempio, ho sempre detto e continuo a ripetere che sono per le maggioranze politiche, ma maggioranza politica

Chi lo sa? Vedremo, ci sarà una legge. Chi la fa questa legge? Il problema è che c'è un *vulnus* che mette in discussione la democrazia. Questo è un fatto molto rilevante. Insisto chiedere al Governo e al Primo Ministro di questo Paese di rispondere a queste domande, perché questo è un problema di democrazia e voi dovete dare una risposta su questo terreno.

alla scelta del Governo di relegare il Parlamento ad un semplice passacarte del potere esecutivo, perché ci si limiterà semplicemente a premere un bottone, senza poter esprimere un dissenso o una valutazione differente rispetto ai provvedimenti del Governo. Ne prendo atto, perché già in legge di bilancio abbiamo visto la maggioranza rinunciare a emendare il testo della legge stessa. Sempre per suo tramite, Presidente, ho necessità di fare una domanda alla ministra Alberti Casellati qui presente, se magari la Ministra presta un attimo attenzione. Vorrei da lei una risposta chiara, una volta per tutte, e non per slogan. Vorrei sapere dalla Ministra se è realmente convinta di sottoscrivere un disegno di legge che non è altro che un furto con destrezza di democrazia. Ministra, ce lo dica per favore, grazie.

vorrei intervenire per fare insieme a voi una riflessione. Accolgo con favore le parole dei colleghi che mi hanno preceduto sul disinteresse generale di questa Assemblea nell'ambito della riforma che invece stessa Assemblea sta portando avanti. Stiamo parlando di una riforma che sostanzialmente fuori, ai cittadini, non interessa granché. Abbiamo visto anche il dato di partecipazione alle ultime elezioni europee,

su una categoria molto importante di astenuti, i giovani, che ad oggi si sentono molto distaccati da questi discorsi che noi opposizioni sostanzialmente facciamo esclusivamente tra di noi,

le vostre riforme vengano prese e smantellate. Voglio ricordare, su tutte, una riforma che ha avuto il consenso la trasversale di tutta l'Assemblea. Lei, Ministra, se lo ricorderà bene (per suo tramite, Presidente). all'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, anche nell'interesse delle future generazioni.

Se non ci riusciamo noi, questa riforma passerà nelle mani dei cittadini, che oggi si sono astenuti, ma nel momento del *referendum* useranno la loro matita per dare un chiaro segno e mettere non una croce come voto, ma proprio una croce su questo tipo di riforma che sta davvero mortificando sia le Assemblee parlamentari che tutto il contesto costituzionale, cui fortunatamente abbiamo il privilegio di poterci appellare. ai nostri Padri costituenti e a tutti i costituzionalisti che si sono espressi su questa riforma. Ecco, noi vi stiamo chiedendo di rifletterci e di pensare. Ministra, ripensi a quei momenti di trasversalità sulle riforme costituzionali già realizzate e guardi quel momento paragonandolo ad oggi e mi dica lei qual è il risultato che state ottenendo.

al Governo, tramite la ministra Alberti Casellati, la domanda delle domande a cui finora non abbiamo avuto alcuna risposta. Sappiamo che cosa pensa il Governo. Quel che sappiamo ci fa paura, ma vorremmo che il Governo uscisse dall'ambiguità e fosse esplicito.

mondiale di un Presidente del Consiglio eletto direttamente, anche l'anomalia non democratica di un Presidente del Consiglio eletto a minoranza e dotato di un potere molto grande come quello che questa riforma gli conferisce? Avete idea di far eleggere il Presidente del Consiglio direttamente dal popolo con una soglia inferiore al 50 per cento e quindi alla maggioranza assoluta? Questa cosa noi dovremmo saperla prima che questo dibattito si concluda, perché non dircela è una grandissima mancanza di rispetto non soltanto delle più elementari regole democratiche (ricordo infatti che in tutti i Paesi dove si elegge direttamente un Presidente, la regola della maggioranza assoluta non conosce eccezioni), ma è anche una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento che si trova a giudicare questa riforma nell'ignoranza rispetto a uno dei suoi punti fondamentali. In questo intervento vorrei lanciare un avvertimento al Governo e alla ministra Alberti Casellati. Ho letto alcune dichiarazioni secondo le quali una soglia del 40 per cento per eleggere direttamente una carica monocratica nazionale sarebbe coperta e legittimata dalle sentenze della Corte costituzionale riguardanti la legge elettorale del 2015. Mi riferisco alla sentenza del 2017. Vi dobbiamo dire da subito che questa è una falsità e una presa in giro. La sentenza della Corte costituzionale del 2017 riguardava la soglia ammissibile per dare un premio di maggioranza per comporre un organo collegiale rappresentativo e non ha niente a che vedere con la soglia che serve per eleggere un organo esecutivo monocratico. Se il Governo non ha la capacità e non ha la voglia di distinguere tra un organo collegiale rappresentativo e un organo monocratico esecutivo vuol dire che siamo messi molto male e, quindi, per amore del Paese e anche per rispetto del Parlamento, la invitiamo a fare chiarezza. Lei vuole un *Premier* eletto dal popolo a colpi di minoranza o è disposta ad accettare

perché non si consumi in quest'Aula un silenzio così triste, così avvilente, sull'articolo che rappresenta il cuore della riforma. Relatore, signora Ministra, prendete la parola, non perché lo chiede l'opposizione, ma per lasciare agli atti per lasciare agli atti di questo Parlamento le vostre considerazioni su come garantire l'attuazione dell'articolo 5 per chi prenderà in mano i Resoconti di questo dibattito e si chiederà come i proponenti, il Governo e il relatore pensano di garantire la maggioranza assoluta dei seggi alle liste collegate e al tempo stesso garantire che non si verifichi l'ipotesi

a chi pensa che questa sia un'Aula di discussione, di confronto. Non vi sembra tristissimo questo silenzio e questo totale spregio nei confronti degli argomenti che abbiamo presentato? Che modo è di riformare la Costituzione?

al proprio interno, tra i deputati e i senatori della stessa maggioranza, un'articolazione di posizione, un dibattito molto acceso. È agli atti, andateli a leggere, e troverete quanti deputati e quanti senatori della maggioranza che sosteneva la riforma sono intervenuti per criticarla, per fare osservazioni, per proporre cambiamenti, presentando emendamenti. In questo caso non c'è niente: il silenzio. Questo è peggio di una anticipazione della riforma che volete approvare.

dicano una parola precisa su questo punto, che è troppo importante, perlomeno per non restare agli atti. In questa sede si sta approvando e si sta l'esame dell'articolo 5, quindi il cuore di questo provvedimento, la settimana prossima faremo le dichiarazioni di voto e avremo finito, il testo passerà all'altro ramo del Parlamento, lasciando quest'Aula e il Paese all'oscuro di questo punto decisivo punto decisivo che riguarda le regole democratiche con le quali si intende mettere a punto la riforma del premierato. È come se noi votassimo una cosa di cui conosciamo il titolo, ma non il contenuto: sappiamo che il Presidente del Consiglio sarà eletto dal popolo, ma incredibilmente non sappiamo come: non sappiamo quanti voti serviranno per eleggere il Presidente del Consiglio, non sappiamo quanto sarà grande il premio di maggioranza, non sappiamo se si intende rispettare la sentenza della Corte costituzionale. Anche nei confronti della Corte costituzionale e degli organismi di garanzia, volete dire una parola chiara su questo o davvero pensate che aver vinto le ultime elezioni vi consenta di esercitare la forza senza però dare alla ragione quella cosa che invece le spetta? Penso che su questo dobbiate dirci delle parole chiare, che dobbiate dirci perlomeno come pensate che debba essere eletto il futuro Presidente del Consiglio e come pensate che debba essere eletto il futuro Parlamento. Non è davvero ammissibile che si concluda la prima lettura

- ve l'ho detto anche prima - un elemento di trasparenza che dovete non semplicemente a noi, ma al Paese, ai cittadini che sono andati a votare, a quelli che non ci sono andati, a tutti a tutti coloro che però pensano giustamente di vivere ancora in una democrazia e che vogliono per l'appunto sapere le regole democratiche di cui si sta discutendo in quest'Aula quali sono oggi e soprattutto quali saranno domani.

Signor Presidente, sono un po' sconcertata dal fatto che ci avviamo a concludere queste votazioni con pochissime dichiarazioni da parte dei dei membri della maggioranza e quelle poche che sono state fatte erano anche sbagliate nel merito di quello che sostenevano, come abbiamo avuto modo di rimarcare diverse volte già ieri e stamattina. Mi domando chi si appresta a votare questo provvedimento che concetto abbia della democrazia o, meglio, se abbia qualche concetto e concezione della democrazia, visto quello che ci che vi assumete la responsabilità di votare e di consegnare al futuro del Paese. Non vi rendete conto di quello che state facendo o forse qualcuno lo vede benissimo. Qualcuno è un utile burattino nelle mani di altri.

lingua italiana e non costituiscono un insulto. Non ho detto "siete dei", ma ho detto "qualcuno è". Signor Presidente, mi interrompa se sbaglio. ritengo di poter argomentare la mia dichiarazione come meglio credo, se non uso insulti

ci siamo sentiti spesso dire, nelle scorse settimane di campagna elettorale, che tanti non vanno a votare, cosa che vi fa sicuramente comodo, perché siamo tutti uguali. Io, invece, oggi lo voglio dire con forza: non siamo tutti uguali! Non lo siamo per niente! E dovreste dirlo anche voi più spesso. Così, quelli che sono stati a casa, cento di italiani che non è andato a votare perché pensa che siamo tutti uguali, forse avrebbe le idee più chiare su chi difende i propri diritti, i diritti dei cittadini italiani e la democrazia, e su chi, invece, aspira solo a ritornare a ritornare ai "fasti" di un ventennio che ci ha portato in una guerra che ha aumentato le divisioni. Una guerra razzista, una guerra che puntava il dito contro quelli che, secondo loro, erano diversi. In quel momento, magari, erano gli ebrei, gli omosessuali e oggi sono individui di altre parti del mondo e altri cittadini, che hanno invece pari dignità, uguale alla nostra. Questo abbiamo scritto nei primi articoli di quella Costituzione che questa maggioranza si appresta a calpestare biecamente. Per questo, noi continuiamo a votare a favore degli emendamenti che la Costituzione vogliono difenderla e voteremo contro questo questo provvedimento che ne vuole fare scempio. Per questo, io ripeto: non siamo tutti uguali! E lo ripeto orgogliosamente.

Signor Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, io non credo che un provvedimento di un Governo possa e debba essere mosso dal rancore, da un sentimento - anzi, un risentimento - di vendetta che schiuma da ogni singolo articolo della vostra riforma (sapete che stento a chiamarla così).

con una gradualità e un lavoro di confronto, secondo un'intenzione equilibrata, ponderata, senza strappi o fughe in avanti, senza la dismisura di una volontà padronale: si fa come dico io o come mi conviene. È esattamente questo il motivo per il quale, la vostra - lo dico tramite lei, Presidente - non è una riforma, ma un tentativo di cancellazione, una *damnatio memoriae*, un regolamento di conti con una Costituzione che non avete mai sentito vostra: una volta preso il potere, finalmente possiamo vendicarci di una Carta che viene da una storia che non riconosciamo, che non sentiamo nostra, che ogni volta ci si pone davanti *(Applausi)* come uno specchio che ci svela, ci denuda, ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. La Costituzione italiana, nella coerenza e nella limpidezza del suo profilo antifascista, è l'antidoto a questo richiamo identitario, proprio perché sradica le appartenenze e le porta sul piano del confronto tra i cittadini, del comune richiamo al gioco democratico, alla difesa delle libertà di ognuno. Libertà, Presidente, che è l'unica vera, profonda, autentica identità degli italiani. Parlando l'altro giorno, in occasione delle commemorazioni per la morte di Giacomo Matteotti, il Presidente della Repubblica ricordava che il coraggio che animò la sua ultima, drammatica denuncia dai banchi di Montecitorio costituisce un atto di fedeltà al Parlamento. Proseguiva il Presidente della Repubblica: «Quel Parlamento che costituisce il cuore di ogni democrazia viva e che venne umiliato dal regime, sino alla sua soppressione». Il cuore di ogni democrazia viva, questo Parlamento, questo Senato, quest'Aula, che di nuovo oggi è sotto attacco. Lo sa, Presidente, che quell'ultimo discorso, quello del 30 maggio del 1924, non fu l'ultima occasione di Matteotti a Montecitorio? Il 4 giugno, appena sei giorni prima del suo sequestro, Matteotti prende la parola in Aula per fatto personale, polemizzando con un deputato, Barbiellini Amidei (un fascista piacentino eretico e incendiario), in una seduta tumultuosa, tanto tumultuosa che a un certo punto lo stesso Mussolini, Presidente del Consiglio presente in Aula, chiese di parlare, dicendo: «Durante il discorso dell'onorevole Facchinetti l'onorevole Matteotti ha accennato a certi atteggiamenti che avrebbe preso il "Popolo d'Italia" durante il 1919. Quali essi siano questi atteggiamenti, io ne rivendico intera la responsabilità; ma io temo che l'onorevole Matteotti mi voglia giocare un brutto tiro, che consisterebbe nel riesumare i discorsi violentissimi che io ho pronunciato, in svariate occasioni, contro l'amnistia ai disertori, discorsi sui quali forse andavano oltre certi certi limiti, che oggi non potrei, per debito di coscienza, mantenere». Matteotti replica e ne nasce un vivace alterco tra i due, con Mussolini mai tanto minaccioso. Dice Matteotti: «Ho ascoltato volentieri le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla questione del decreto di amnistia ai disertori. Trovo in esse una leale accettazione del fatto che io ho enunciato». Mussolini: «Dimostrerò il contrario». Matteotti: «L'apprezzamento di quelle frasi stampate nel 1919 sul "Popolo d'Italia" può essere poi fatto dal pubblico. Noi abbiamo pubblicato sul nostro giornale il testo». Mussolini: «Non i miei discorsi». E Matteotti replica: «Non vorrà certo che noi pubblichiamo l'edizione completa dei suoi lavori!». Mussolini: «Lo fate tanto spesso! Vivete ancora su quello. Riportate sempre i miei articoli dopo dieci anni. Persino il 1° maggio!». E Matteotti: «Abbiamo pubblicato solamente, si intende, la parte che ci interessava come avversari e cioè l'approvazione dell'amnistia, data nel vostro giornale nel febbraio e nel settembre del 1919. Le pubblicazioni restano non smentibili; e ognuno ha i suoi errori, sui quali poi il pubblico formula il suo apprezzamento. Perciò questo incidente è chiaramente liquidato!». «Io dimostrerò la vostra mala fede». A quel punto prende la parola Barbiellini Amidei, che in questo clima lugubre polemizza e ironizza su Matteotti e gli dice:

gridando: «A me no!». Queste tre parole sono le ultime effettive che Matteotti pronuncia in Parlamento: "a me no". Si riferivano ad altro, come avete sentito, ma mi sono parse una sintesi perfetta della resistenza strenua di Matteotti al fascismo e della sua radicale assoluta alterità a Mussolini.

della sua forza di opporsi agli abusi, all'arroganza e alla violenza, con gli strumenti della democrazia, con il rispetto delle regole e con la difesa del Parlamento che, ieri come oggi, resta

Signor Presidente, Ministra, colleghi, se provassimo a guardarci da fuori, non pensando di essere seduti su questi scranni, credo che l'impressione sarebbe quella di lunghi monologhi che non trovano alcuna risposta. Mettiamoci nei panni di chi ci guarda nel Paese.

difficili da non rendere possibile la discussione. E invece no. Noi stiamo discutendo della vita democratica del Paese e di ciò che poi, alla fine, condiziona la vita, la libertà e le scelte di ogni singolo cittadino o cittadina di questo Paese. Ed è davvero intollerabile che tutto questo avvenga senza che ci siano le risposte che ci permettono anche di giudicare quello che stiamo facendo: come voteremo, come decideremo la nostra rappresentanza, quali poteri effettivi avrà un Parlamento che, come abbiamo detto tante volte, viene eletto a strascico, come sarà possibile garantire quell'equilibrio di poteri che impedisce a un singolo di determinare il destino di tutti senza alcun confronto democratico. Ciò non vi sollecita alcuna pulsione e necessità di provare a interloquire, nessuna volontà di provare a spiegare ai cittadini di che cosa stiamo discutendo. Voi forse immaginate che ciò possa rappresentare la vostra prova di forza comunque andare avanti), mentre ciò che lascerà sarà il segnale che questo Parlamento non rappresenta il Paese e non è in grado di interloquire con esso. Credo che convenga anzitutto alla maggioranza essere in grado di dire che cosa vuol fare davvero e dare delle risposte, perché il non farlo rappresenterà solo un altro grande argomento, per noi, affinché questa non diventi la riforma del Paese.

perché diciassette sono le ore che non vengono utilizzate dalla maggioranza per intervenire. Quando si dice che interverremo per trenta ore non è vero. E perché la maggioranza non interviene? È un anticipo di premierato, esattamente quello che succederà quando questa riforma sarà approvata con il *referendum* dagli italiani (cosa che io mi auguro non accada). In un ipotetico futuro in cui ciò avvenisse, la maggioranza sarà costretta a questo.

un solo collega di maggioranza difenda questa riforma. Al netto di quanto si fa apparire esternamente, nell'intimità di queste stanze ogni singolo membro di questa maggioranza, di qualsiasi forza politica, esprime enormi perplessità su questo testo. È un testo che si basa su alcuni assurdi. Vi sono presupposti su cui tutti noi concordiamo: la governabilità, il

vi è stata una tornata elettorale in cui c'è stato un voto di preferenza per Giorgia, che ha avuto un enorme successo elettorale, riconosciuto da tutti. quindi lecito pensare che questa maggioranza, che ha avuto un successo elettorale, sarà quella che potenzialmente domani, a elezioni politiche a Costituzione vigente, porterà a casa il risultato della vittoria: Giorgia sarà di nuovo Presidente del Consiglio. Ma ci sono delle forze politiche che sono determinanti per la maggioranza; se una di queste, ad esempio la Lega, che magari non vede approvata l'autonomia differenziata, decide di togliere la fiducia Giorgia, a un incarico, magari a uno dei Vice Presidenti del Consiglio, magari a Matteo, che magari avrà la maggioranza con tutto il resto del Parlamento. E quello non sarà un inciucio possibile con questa nuova Costituzione? Certo che lo sarà. Ma se poi magari Matteo ha un impedimento, non esiste più una possibilità per il Parlamento, perché dal secondo Presidente incaricato in poi il Parlamento muore, così, senza motivazioni politiche, per un un'eutanasia costituzionale. Questa è una riforma assurda della Costituzione e, nell'intimità di queste stanze (non di quest'Aula, ma nelle stanze qui dietro), tutti lo state dicendo. Stiamo allora parlando del nulla. *(Applausi)*. Questa riforma non è quella che verrà portata a termine. Se c'è bisogno di eutanasia, serve a questo testo e non alla nostra bellissima Costituzione. solo per aggiungere qualche riflessione a quelle che faceva ora il collega Patuanelli, che secondo me ha detto parole molto giuste, molto corrette, anche rappresentando questa discussione, come

alle ultime battute, su un provvedimento di prima grandezza, ossia la riforma costituzionale, quindi non un provvedimento che si fa tutti i giorni, un semplice decreto-legge in scadenza, ma una delle norme più significative e più importanti

Si vede proprio in questa discussione, con le forze di opposizione quasi messe in una condizione di impotenza e i parlamentari di maggioranza che rinunciano alle diciassette ore citate dal collega Patuanelli sul totale delle trenta complessive destinate a questo dibattito. Già ora, in questa discussione, si vede come tutto quello che è successo in tutti questi anni abbia, finanche psicologicamente, non semplicemente formalmente, messo il Parlamento in una condizione di difficoltà. Guardate che la discussione di questa settimana è molto indicativa ed è proprio la dimostrazione di come trent'anni di indirizzo politico-culturale portato avanti in un certo modo (il leaderismo, il maggioritario, il partito del capo, i premi di maggioranza, tutto quello che è successo in questi trent'anni) già oggi, a Costituzione vigente, quindi prima della riforma del premierato, hanno modificato l'atteggiamento che invece un tempo aveva segnato le pagine più belle della storia di questo Parlamento. Quanto sono lontane da questo dibattito che stiamo vedendo ora quelle pagine gloriose fatte in tempi passati, quando invece la vita democratica, il radicamento dei partiti, le discussioni, anche le più aspre in quest'Aula, erano però la testimonianza di partiti che avevano una connessione reale con la società civile vera di questo Paese, che portavano avanti e rappresentavano pezzi di interesse, con questa parola considerando le ragioni più nobili. Penso che tutto questo avrebbe dovuto essere al centro di questa discussione; invece è stato tirato via. Noi stiamo discutendo di come cambiare la Costituzione italiana su un punto essenziale, facendo finta che questi trent'anni non ci siano stati, facendo finta che non abbiamo a che fare con un progressivo svuotamento dell'istituzione democratica massima di questo Paese e anche il dibattito di queste settimane drammaticamente lo dimostra. Di questo avremmo avuto bisogno: discutere di come intervenire e come migliorare, per l'appunto, il Parlamento repubblicano. Cosa andiamo a fare invece? In una condizione già di grande sofferenza come questa, con questo spettacolo che stiamo dando all'esterno di un Parlamento muto

riforma - se ci riuscirete, ma io ve l'ho detto tante volte, sono convinto che alla fine non sarà così, perché la saggezza del popolo italiano sarà molto più grande di chi invece li rappresenta (male) dentro quest'Aula *(Applausi)* -, se malauguratamente questa riforma dovesse vedere la luce, questi aspetti vedranno ulteriori elementi di torsione. È questo il vero elemento di grande preoccupazione. Ma davvero ci possiamo rassegnare a un Paese in cui l'istituzione massima della Repubblica venga così clamorosamente messa da parte? Davvero possiamo rassegnarci all'idea di dover eleggere quelli che verranno dopo di noi per trascinamento, semplicemente perché fanno parte di liste collegate al Presidente del Consiglio, peraltro probabilmente senza la maggioranza dei voti, con premi di maggioranza abnormi, quando mezzo Paese, se va bene, guarderà questo spettacolo in televisione, senza nemmeno voler partecipare al gioco democratico? Nel frattempo, infatti, come sta accadendo ogni elezione che passa, si abbassa sempre di più la percentuale di quelli che vanno al voto. Le avete viste le percentuali di tutti i nostri partiti, depurate dall'astensione? Guardatele le percentuali di tutti i nostri partiti depurate dall'astensione e scoprirete che il 29 per cento di Fratelli d'Italia diventa il 15 cento e naturalmente, a cascata, i voti di tutti gli altri; finanche un risultato significativo come quello che ha preso il mio partito dimezza, com'è evidente, quando si misura il fatto che mezzo Paese non va più a votare. Li avete visti questi dati, oppure non vi dicono niente? Vi volete misurare con questa realtà, oppure fate finta che non c'è, che non esiste? esiste? *(Applausi)*. Per questo ieri dicevo che dovremmo mettere un cartello là fuori con scritto «chiuso per lutto» dinanzi a questo disastro che sta accadendo in Italia, peraltro dinanzi al fatto che questa astensione cresce di più dov'è più acuta la sofferenza sociale, al Sud, nei quartieri più periferici, nei quartieri più poveri, dove non va a votare più nessuno. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme gigantesco per tutti quanti noi. Invece cosa si fa dinanzi a questa crisi democratica così clamorosa? Si sceglie di accentuare la crisi democratica, si sceglie una strada scorciatoia che questo distacco tra la popolazione, i partiti e le istituzioni inevitabilmente accentuerà. Si sceglie per l'appunto una strada che sarà - io credo - molto pericolosa per la nostra democrazia. Siamo ancora in tempo. Ve lo dico per l'ultima volta: fermatevi, anche sulla base di quello che è successo domenica scorsa, facciamo i conti con questa realtà di cui ci parla un Paese reale, un Paese in sofferenza. Ce lo stanno dicendo in tutti i modi; non facciamo finta di niente, cerchiamo di rispondere a questo tipo di domanda l'appunto, a fare un dibattito all'altezza di quello che servirebbe al Paese e non invece alla propaganda che si sta facendo da molti mesi in quest'Aula parlamentare.

Quando, durante l'approvazione dell'autonomia differenziata, che purtroppo è al voto finale alla Camera, in Commissione bilancio abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva sui profili finanziari di quella legge (che, ricordo, non è stata incardinata in Commissione bilancio), l'abbiamo fatto perché c'erano l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Commissione europea e Bankitalia che ci dicevano di fare attenzione a permettere alle Regioni di trattenere il gettito fiscale, perché ciò vuol dire che ci saranno meno risorse a disposizione delle Regioni più povere e che i divari che ci sono oggi non potranno che aumentare in questo assetto. Chiedevamo quell'approfondimento e ancora lo chiediamo, perché siamo convinti che quella legge, senza aver chiarito quei profili finanziari,

prima di approvare l'articolo 5, si deve chiarire qual è la legge elettorale che si vuole fare, lo facciamo perché siamo convinti che quello che è stato detto in audizione sia pericoloso, cioè senza dire qual è il premio di maggioranza e come si vuole fare in modo che il *Premier* traini con sé anche il Parlamento. È un sistema che non esiste da nessuna parte al mondo, e ci sarà un motivo. Se anche dove è stato sperimentato il premierato c'era un Parlamento eletto separatamente, ci sarà un motivo. Vede, Presidente, ci dicono che c'è una maggioranza che vuole collaborare e un'opposizione che invece pensa a fare l'opposizione e non entra nel merito della questione. Vorrei ricordare che la mia forza politica ha presentato una manciata di emendamenti, che si contavano sulle dita di una mano. Erano Erano emendamenti che davvero miravano a rendere più stabile il Governo: c'era la sfiducia costruttiva, c'era la fiducia a Camere riunite, c'era la possibilità

il presidente Patuanelli. C'è un secondo *Premier* che ha quasi più poteri del primo, tanto che avete dovuto apportare dei correttivi. Avete addirittura scritto che poteva essere resuscitato il primo *Premier*, a cui poteva essere nuovamente conferita la fiducia. Ci sono degli errori madornali in questa legge, che vi abbiamo chiesto di modificare nel merito. Ma anche qui scena muta. Non abbiamo capito in che modo volete risolvere questi problemi. Lo dico di nuovo alla Ministra e al relatore: fateci capire come intendete superare i problemi di merito che ci sono in questo testo, anche nell'articolo 5. La campagna elettorale è finita, la propaganda si deve chiudere. Qui abbiamo una Costituzione che state distruggendo. *(Applausi)*. State alterando gli equilibri costituzionali, senza dire in che modo volete mettere dei correttivi. Questo è il momento di dirci come lo volete fare. Avete fatto addirittura campagna elettorale sulla pelle delle persone e dei malati, annunciando e approvando un decreto liste d'attesa, che ha le liste d'attesa solo nel titolo, a costo zero, anche quello. Non c'è un euro per l'assunzione di personale sanitario *(Applausi)* che sappiamo essere l'unica cosa che davvero serve per accorciare le liste di attesa. di attesa. Dimostrate, in conclusione, di essere patrioti come vi professate, difendete il Paese anche quei cittadini del Sud che hanno deciso di non andare a votare perché ormai non credono più che le istituzioni possano in alcun modo tutelarli, sono disperati,

Diventate patrioti e fateci capire anche in quest'Aula in che modo siete patrioti e come volete difendere la Costituzione.

vice presidente Castellone, che è esattamente la prosecuzione di quello che le colleghe e i colleghi hanno detto sull'articolo 5. Mi rivolgo ai Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza: fermatevi fin quando siete in tempo. Signora Presidente, siamo molto preoccupati perché prima delle elezioni europee c'era una luce di speranza nonostante alcune cose che non condividevamo. C'era ad esempio il presidente Pera che interveniva sulla Britannia, ora evidentemente è stato colto dalle riflessioni fatte sulla monarchia e anche lui ha perso la parola. C'era l'energia un po' repressa, ma sempre viva del collega Menia, ma vediamo che non interviene più nemmeno lui. C'era il presidente Balboni che in qualche modo ogni tanto reagiva alle nostre richieste e provava a dirci qual era la speranza - a questo punto vana - che la maggioranza aveva. Soprattutto gli appunti della ministra Alberti Casellati si trasformavano in alcune risposte; molte, le devo dire, non ci convincevano, ma almeno ci provava. Oggi silenzio assordante. Quello che non capiamo è se il silenzio è obbedienza o una libera scelta dei colleghi di maggioranza. Noi temiamo che sia semplicemente obbedienza. *(Applausi)*.

siano le prove generali rispetto ad un premierato che noi abbiamo contestato dal primo momento non perché non cogliessimo il tentativo di provare a modificare la Costituzione,

oppure sono imbavagliato? PRESIDENTE. Le sto dando tutto il tempo che vuole. BOCCIA *(PD-IDP)*. In tutto questo, signora Presidente, i tempi larghi a disposizione della maggioranza non sono i tempi che ha l'opposizione. L'opposizione ha provato a far cambiare tesi e valutazioni, a spingere la maggioranza verso un confronto di merito che non riguarda un disegno di legge di una senatrice o di un senatore dell'opposizione, ma la nostra Costituzione. La Costituzione che ricorda sempre quest'Aula e che ricordano quanto lei si ritrova dietro le spalle ogni volta che presiede, le parole solenni che sono scolpite sulla parete.

la vita del Paese e il funzionamento della nostra democrazia. Prendiamo atto che la nostra richiesta di maggior tempo non è stata ancora esaudita, perché, pur parlando a spizzichi e bocconi, tra un emendamento e l'altro, di fatto non siamo in grado di valutare i tempi che abbiamo a disposizione e quindi quale sforzo dobbiamo fare sugli altri articoli di questa pessima riforma. Per queste ragioni,

si pensa di approvare un articolo con cui si interviene sulla questione della forma di governo e della forma della forma parlamentare, però senza dire esattamente in quale direzione si vuole andare. Abbiamo cercato di spiegare

discriminazione, non sono per niente rappresentate. Guardiamo alla composizione di questo Parlamento, sia al Senato sia alla Camera: ci sono molte fasce di cittadini che non sono rappresentate,

Allora discutiamo di questo e vediamo come fare, ad esempio stabilendo regole democratiche. Penso, ad esempio, che bisognerebbe ripristinare il ruolo e anche il finanziamento dei partiti, togliendo magari ai singoli deputati e senatori,

Adesso la questione dei cambiamenti dei Gruppi parlamentari è già diversa, però in passato, fino al passato recente, era molto più facile. Chi ti elegge, chi ti ha portato in Parlamento, rischia di non avere più nessuna risorsa perché chi è eletto ha cambiato opinione. È possibile cambiare opinione, ma chi ti ha eletto deve continuare a godere del voto che ha dato a un determinato partito. Vogliamo discutere di questo? Vogliamo discutere di un problema di rappresentanza sociale? Anche fuori dal Parlamento c'è un problema di rappresentanza.

che il sindaco d'Italia, come qualcuno lo aveva definito, risolva i problemi? Normalmente i sindaci non fanno le leggi, ma sono esecutori di leggi che fa il Parlamento, quindi dobbiamo distinguere tra questione esecutiva e questione

Signor Presidente, faccio mie le inquietudini della collega, senatrice Camusso. Com'è possibile che una riforma di così vasta portata, che incide in profondità sulle libertà fondamentali del cittadino, passi in questo modo, che definire surreale è un eufemismo? passando in un contesto costellato dal silenzio della maggioranza, che si sottrae al dibattito e al confronto, e nell'assordante silenzio del Governo che, soltanto da estemporanee dichiarazioni di stampa, sappiamo aver detto che questa è una riformetta che praticamente incide su una manciata di articoli della Costituzione. In sostanza, che volete che sia! Come se contasse il numero degli articoli modificati, anziché la sostanza delle modifiche apportate al testo della Costituzione. *(Applausi)*. Sappiamo invece che anche un frammento di norma, se incide sulla sostanza dei rapporti, può essere devastante. Siamo qui in presenza di un meccanismo veramente terrificante. Sono convinto che la stessa maggioranza non sia consapevole non sia consapevole di cosa si stia facendo. Qui si sta sostituendo a un sistema costituzionale nettamente fondato sulla divisione dei poteri, sui ruoli distinti dell'esecutivo e del legislativo e sul ruolo di garanzia del Capo dello Stato, un sistema pasticciato, un ircocervo giuridico, un sistema che Giovanni Sartori avrebbe definito senza né capo, né coda, un bi-presidenzialismo zoppo e claudicante in cui il Capo dello Stato viene ridotto a un simulacro. Altro che Altro che organo di garanzia, di cui ci sarebbe oggi una necessità molto più forte che in altre epoche storiche! Sta infatti passando la riforma spacca-Italia, che divide in due il Paese, in cui l'unica possibilità ancora di riconoscersi in una unitarietà di valori e ontologica è nelle mani del Capo dello Stato. Se però costui è indebolito e neutralizzato in questa funzione, capiamo bene che rimangono l'Italia divisa in due e un Presidente della Repubblica che è il simulacro di un Capo dello Stato. Questa è una riforma pasticciata, che inverte completamente l'ordine dei rapporti disegnati nella Costituzione; è un nuovo modello costituzionale affatto antitetico rispetto a quello originario, che sta passando in queste forme surreali di cui abbiamo detto. Invito la maggioranza ad andarsi a leggere - o a rileggere, per chi già la conoscesse - la parabola del leone di Eschilo, del leone di Eschilo, che, quando era un piccolo leoncino, era il trastullo del re; quando divenne grande, lo divorò. Voi state costruendo un sistema del quale potreste essere vittime e non siete consapevoli di cosa vi state facendo.

domani, in base ai corsi e ricorsi che Giambattista Vico ci ha insegnato appartenere al necessario fluttuare della storia, potreste essere nella condizione di subire l'assalto dell'ircocervo

*do ut facias*), nella doppia accezione del termine, come descritto dal Devoto-Oli, dizionario della lingua italiana: come accordo furbesco e fraudolento, spregiudicato e mercimonioso, e come pasticcio. Noi vi esortiamo e mi ricollego alle esortazioni del nostro capogruppo Patuanelli e del senatore Boccia: fermatevi, siete ancora in tempo. Ma non Ma non sentite, nel fondo della vostra coscienza, la necessità di recuperare un sussulto di dignitosa coerenza? Voi siete quelli che il 22 agosto hanno sottoposto all'elettorato un programma di governo, firmato da tutti quanti voi, in cui si proponeva l'elezione diretta e popolare del Presidente della Repubblica. State cambiando le carte in tavola, frodando dapprima i vostri elettori e poi tutto il popolo italiano. *(Applausi)*. Recuperate la dignità e la coerenza, siamo ancora in tempo. siamo ancora in tempo. Vi esorto poi ad avere maggiore rispetto per il Parlamento di cui fate parte.

La prego di concludere, è al settimo minuto. CASTIELLO *(M5S)*. Pensate a quello che dice e prescrive la Corte costituzionale, con statuizione chiara e certa: la compromissione dei poteri del Parlamento...

la frammentazione partitica e l'instabilità dei Governi. Tuttavia, non possiamo dimenticare che, nonostante il ricorso a leggi elettorali maggioritarie, la frammentazione partitica sia proseguita e la bipolarizzazione coatta del sistema politico non abbia affatto reso più stabili i Governi, né quelli di centrodestra, né quelli di centrosinistra. a questi tentativi - naufragati - di utilizzare la riforma della legge elettorale per produrre stabilità e superare la frammentazione, oggi ripartiamo da capo, come se nulla fosse successo, con un sistema che addirittura costituzionalizza la legge elettorale e determina l'elezione diretta del *Premier*, una legge elettorale senza una soglia definita, quindi con un'anomalia ancora più forte rispetto ai tentativi di riforma che già in passato non hanno dato risultati. risultati. Oggi voglio confermare la linea di Azione, ovvero il convincimento che l'elezione diretta del Capo dell'Esecutivo, con la contestuale definizione degli stessi poteri precedentemente vigenti, senza un adeguato rafforzamento, non sia la strada per rendere più stabili gli Esecutivi. L'elezione del Capo dell'Esecutivo può determinare un rafforzamento, laddove si rafforzino anche i poteri e le competenze, ci sia un adeguato ruolo del Parlamento e la legge elettorale non sia contenuta all'interno della Costituzione, ma venga prevista una soglia minima. Così, con questo sistema, noi riteniamo che la soluzione non solo non stabilizzi i Governi, ma determini la stessa frammentazione che abbiamo vissuto fino ad oggi. Ecco perché, secondo noi, questo articolo è profondamente da rivedere. La ringrazio,

che poi sono sempre le stesse, anche in merito all'articolo 5 della legge elettorale, hanno avuto puntuale risposta, sia in tutto il dibattito che c'è stato in Commissione, sia in alcuni interventi che la maggioranza ha fatto in quest'Aula, sia nella risposta del Ministro, sia nella risposta del relatore. Anche quando accompagno mia figlia da qualche parte, appena ci sediamo in macchina mi chiede «tra quanto arriviamo?»,

particolarmente spiacevole che quando è intervenuto il Ministro, facendo una lunga relazione, molti di voi fossero distratti, al telefono, facessero completamente altro e non l'ascoltassero, perché, come vi dicevo, la risposta sulla legge elettorale è molto banalmente che, se questa maggioranza avesse presentato una riforma costituzionale affiancata a una legge elettorale, avrebbe voluto dire che il Parlamento era completamente mortificato, perché evidentemente la riforma costituzionale sarebbe stata immodificabile. Quella, sì,

le riflessioni delle opposizioni. Vi dico e vi chiedo di più: spiegatemi come sia possibile presentare una legge elettorale su una riforma costituzionale che non è stata ancora approvata. Perché di questo si tratterebbe, cioè di depositare il testo di una legge elettorale che prevede cose sulla base di una Costituzione che ancora non è stata approvata e non è esistente. Mi domando e vi domando come sia possibile e cosa direbbe il Presidente della Repubblica, se si vedesse arrivare una legge che modifica qualcosa che ancora non è stato modificato. Credo francamente che non sia corretto nei confronti né del Parlamento, né di una Costituzione che allo stato degli atti, anche una volta approvato questo testo, non sarebbe ancora stata approvata e molto probabilmente dovrebbe passare anche attraverso un *referendum* da parte del popolo. La legge elettorale, molto banalmente, non poteva e non può essere presentata come affiancata a questa, a maggior ragione nella consapevolezza che il percorso di una legge elettorale e quello di una riforma costituzionale hanno tempi ben diversi. Paradossalmente, ci troveremmo nella condizione di approvare una legge elettorale su una Costituzione che ancora non è stata modificata, quindi era impossibile. Dopodiché, rispetto alle osservazioni che sono state fatte sulla possibile legge elettorale, dicendo che non abbiamo detto niente, anche questa è una falsità e anche questa, nonostante la ripetiate più volte, è inutile. È inutile, molto banalmente, perché non inserire in Costituzione la legge elettorale è una maggiore garanzia per l'Italia e per tutti i pericoli fantomatici che avete manifestato in quest'Aula. Trattandosi infatti di legge subordinata alla Costituzione, la legge elettorale deve rispettare in maniera ancora più rigida e ferrea i principi che saranno dettati nella Costituzione e che sono stati dettati puntualmente dalla stessa Corte costituzionale,

richiamare). La legge elettorale rispetterà tutti i principi che sono stati dettati dalla Corte costituzionale nelle note sentenze che in molti casi sono state richiamate. Saranno totalmente impossibili premi di maggioranza

l'ipotesi del ballottaggio è una possibilità molto concreta, che certo sarà in campo, perché è impossibile conferire un premio di maggioranza superiore al 50 per cento a un partito che ha preso il 25, il 26 o il 30 Quindi le risposte vi sono state date tutte. Dico una cosa molto sommessamente, perché il senatore Sensi prima ha urlato di stalla.

Continueremo ad affrontare con la massima serietà, come abbiamo fatto sinora, questa riforma costituzionale, che è fatta per l'Italia e per gli italiani, che meritano maggiore serietà e rispetto. Grazie.

Sì, è così, non siete il partito più grande, ma io credo che la Presidenza non abbia problemi a darvi comunque questa opportunità. Presidente, la ringrazio di questo ulteriore tempo, ma mi lasci esprimere il rammarico per

Se noi avessimo ascoltato prima queste considerazioni e se ci fosse stata la disponibilità del Governo, del relatore e dello stesso senatore Lisei a a entrare nel merito delle considerazioni che ha svolto, noi avremmo dato dignità a quest'Aula. Avremmo dato un ruolo a questo Parlamento. Il senatore Lisei, che cito

ricorrendo al ballottaggio. Questa risposta se noi fossimo in un'Aula che vuole davvero prendere sul serio il confronto, andrebbe approfondita con tutto il rispetto naturalmente per l'ultimo intervento che ho ascoltato, dire che la legge futura rispetterà i principi della Corte a noi non basta. Vorremmo sapere come li rispetterà. *(Applausi).* Ripeto e ci ritorno sopra

superiore al 51 per cento dei seggi attribuiti, che non corrisponda almeno a un voto per quelle liste superiore al 40 per cento. Si possono fare tutti i ballottaggi che si vogliono, ma quando noi sottolineiamo il problema della disproporzionalità tra il numero dei seggi attribuiti alle liste collegate e il numero di voti conseguiti dalle liste, non ci riferiamo al problema, pur fondamentale anch'esso, di di quanto consenso occorre per legittimare il Presidente del Consiglio, ma di quanto consenso occorre alle liste per avere legittimamente il premio di maggioranza.

per definire le condizioni dell'attribuzione del premio alle liste, che in questo testo costituzionale si prevede che debba scattare necessariamente - perché si dice garantisce - in relazione all'elezione del Presidente del Consiglio. A noi sembra che anche una legge che eventualmente prevedesse il doppio turno per l'elezione del Presidente del Consiglio non risolverebbe il problema del rapporto tra numero di voti ottenuti dalle liste collegate e numero di seggi attribuiti. fossimo consapevoli del ruolo che svolgiamo e anche un po' orgogliosi di svolgerlo, approfondiremmo questo problema, non chiuderemmo il dibattito. Non considereremmo queste nostre argomentazioni come pretestuose ed ostruzionistiche, ma, al contrario, come considerazioni di merito che meritano una risposta. Non c'è niente da fare, da questo problema non si esce ed è il motivo per cui l'articolo 5, al di là della concentrazione inedita di potere e dello stravolgimento della funzione del Parlamento, stando a quello che abbiamo ascoltato dagli auditi e a quello che abbiamo detto, non

di protagonismo. Questo sussulto di protagonismo è possibile però solo se lei riapre i termini *(Applausi)*, rinuncia al contingentamento e ci consente di dialogare, di confrontarci, altrimenti non è possibile

La seduta è sospesa.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ricorre un anno dalla scomparsa del presidente, senatore Silvio Berlusconi, eletto anche in questa legislatura al Senato della Repubblica. La vita di Berlusconi e la sua storia sono parte della storia italiana del nostro tempo, ma voglio, in questa occasione, ricordare soprattutto il tratto umano di Silvio Berlusconi, che, pure con il suo ruolo e con la sua storia, aveva sempre l'umiltà dell'ascolto. La sua cortesia era apprezzata da tutti. Anche con le persone più distanti da lui sapeva avere sempre un approccio gentile. Segnava tutti i pensieri che ascoltava; con il suo tipico pennarello, annotando le discussioni che si svolgevano intorno a lui e che seguiva con attenzione. Dicevo del tratto umano. Nel dicembre del 2009 avevo perso mia madre. Ovviamente, era per me un momento particolare. Suonò il telefono. Era il presidente Berlusconi, che la sera prima - era il dicembre 2009 - aveva ricevuto una statuetta di granito sul volto: un episodio che penso tutti ricorderanno.

che ancora ricordo, sulle mamme, su sua mamma, sulle nostre mamme. Questo è Berlusconi. Cito questo fatto assolutamente personale per ribadire chi sia stato Berlusconi. Le imprese politiche, pubbliche ed economiche, infatti, le conoscono tutti, ma la sua umanità è ciò che noi dobbiamo ricordare più di tutto. È stato primo in ogni cosa che ha fatto. Primo nell'edilizia, con una capacità di edificare modelli a misura d'uomo; un ambientalista del fare e non della demagogia. È stato primo nel calcio, prendendo una squadra, cui era legato, che era in crisi e portandola al vertice mondiale, come lui aveva profetizzato, con interlocutori increduli quando furono chiamati a condividere quell'impresa che sembrava impossibile. È stato primo nelle televisioni, con grandi innovazioni e tante polemiche inutili, perché, come prevedemmo anche in quest'Aula in tempi andati, poi il mercato dell'offerta televisiva si è allargato a dismisura, con tutto quello che nel tempo si è aggiunto. È stato primo nella politica. Nessuno è stato alla guida del Governo per un tempo pari al suo. Ha valorizzato classi dirigenti, ovunque nelle sue aziende. aziende. Recentemente, un docufilm su di lui è stato il più visto, per alcune settimane, su una piattaforma televisiva; così come il libro che Paolo Del Debbio ha dedicato a Silvio Berlusconi, al primo programma di Forza Italia, pubblicando anche alcuni scritti degli ultimi giorni di Berlusconi, con una calligrafia che la malattia rendeva incerta, ma con pensieri chiari, è stato il libro più venduto per alcune settimane. Quindi, l'effetto Berlusconi ancora si propaga nei documentari, nei film, nei libri che di lui parlano. È È stato il primo in tanti contesti. Il presidente Confalonieri ha detto, proprio in questo docufilm, una frase che io ho conservato: l'ho incorniciata e la tengo nel mio ufficio, perché è un monito, per me stesso e per tutti. Dice Confalonieri, che con Berlusconi ha condiviso un'intera vita: noi, con Berlusconi, siamo diventati Presidenti di qui e Presidenti di là. Ma Berlusconi sarebbe stato Berlusconi con altri al posto nostro. Un'affermazione di grande umiltà da parte di Fedele Confalonieri e che propongo a tutti noi, a me stesso per primo, e a noi che abbiamo vissuto l'epopea berlusconiana. Io facevo parte addirittura, come giovane Sottosegretario, del primo Governo Berlusconi del 1994. L'abbiamo vissuta con i nostri limiti, le nostre capacità, ma certamente al di sotto della sua grandezza. Forse questa è una riflessione che in politica, indipendentemente dagli schieramenti, dovremmo fare tutti per richiamare noi stessi all'umiltà. giornalisti, persone nelle televisioni, *manager*, ha creato opportunità di lavoro e di crescita a tantissime donne e uomini. Ha creato spazi per tanti in politica, ha fondato il centrodestra con quella celeberrima "discesa in campo". Ha favorito il bipolarismo, ha messo fine alla palude consociativa, ha dato lavoro perfino a chi ha fatto dell'aggressione incessante alla sua persona una ragione di vita e di guadagno. Alcuni non sarebbero diventati celebri se non avessero avuto l'ossessione di Berlusconi nella loro immutabile agenda polemica. Ha pagato prezzi durissimi accanto alle soddisfazioni enormi, subendo autentiche persecuzioni, ma non è questa oggi l'occasione per parlarne. Oggi ricordiamo l'uomo, la persona, non dobbiamo essere divisivi. Oggi ricordiamo anche il Berlusconi uomo della pace, quello che nel 2002 a Pratica di Mare aveva messo Putin e Bush allo stesso tavolo. Quanto servirebbe oggi al mondo uno statista di quella dimensione, quello che parlava con gli interlocutori più ostici, i Gheddafi e i Putin, perché la pace si mantiene parlando con la gente difficile, più che con i buoni parlando con i cattivi della storia. È quindi un onore, colleghi, oggi parlare, a nome di Forza Italia e del nostro Gruppo. Voglio anche stringermi attorno alla famiglia e ai suoi figli, che hanno dato una dimostrazione esemplare in questi dodici mesi per come hanno saputo gestire una situazione di grande rilievo, una transizione tutt'altro che banale, un esempio virtuoso, evidentemente anche frutto di un grande insegnamento. In conclusione, questa sera in televisione sui canali Mediaset andrà in onda una programmazione speciale, come prevedibile, a un anno dalla scomparsa e Toni Capuozzo, che - ho sentito negli spot - ha curato questo programma, ha detto una frase che evidentemente questa sera sentiremo: Berlusconi è un uomo che ha vissuto troppe vite per morire del tutto. Non saprei usare parole migliori per unirmi a tutti voi nel ricordo di un grande italiano. *(Applausi)*.

del nostro emiciclo, nel ricordo di Silvio Berlusconi, che - come molti in quest'Aula - ho avuto il piacere, vorrei dire l'onore, se non mi correggete, di apprezzare e conoscere. Non voglio parlare dei Ministri che l'hanno conosciuto, credo tutti; cito solo tra i Ministri il ministro degli affari esteri Tajani, che fino alla fine è stato

e tanti altri parlamentari. Non li voglio citare tutti, uno ad uno. Che cosa ha fatto di unico Berlusconi? Io credo che lui avesse veramente non la capacità di sognare, che ce l'hanno in tanti, ma la capacità di realizzare i propri sogni. Lo ha fatto quando è sceso in campo, come diceva lui, perché prima non esisteva questa frase, scendere in campo, semmai si saliva in politica.

e Bossi potessero fare parte della stessa maggioranza. Tant'è vero che dopo, prima che Fini e Bossi tornassero a riprendere un caffè insieme, so io la fatica che ho dovuto fare anche personalmente. Ma in quel momento solo Berlusconi poteva immaginare di creare una coalizione così innovativa, così impossibile anche solo da sognare e immaginare vincente. Non dimenticate che con gli stessi sogni realizzati ha costruito una città che ancora oggi è

un sogno e lui tranquillamente lo realizzava. Chi poteva immaginare che in Italia vi fosse uno spazio per le televisioni private concorrenziale

fallimento, potesse diventare la squadra più titolata del mondo? Lui l'ha detto appena l'ha comprata e l'ha realizzato. Potrei andare avanti con esempi di questo genere, che valgono più di mille parole di circostanze. Poi, certo, è stato un uomo anche molto discusso, un uomo che ha avuto, credo, tanti elogi e tanti amici quanti ne ha avuti di opposti, di avversari, qualche volta di nemici. Ha sempre combattuto la sua battaglia giudiziaria e, comunque la si voglia guardare, anche quella unica nella storia della politica italiana. Berlusconi se n'è andato forse troppo presto, forse nel momento in cui poteva dire: il ciclo adesso lo consegno, perché è un ciclo ancora con i miei sogni vincenti, che era quello di una larga parte politica che esisteva, il centrodestra, solo perché lui l'aveva sognato, immaginato e voluto. Se n'è andato e devo dirvi - stavolta parlo a titolo personale - che ci manca; ci manca anche l'ultimo Berlusconi, quello che era un punto di riferimento. Non era più il partito più grande,

oltre che un ricordo per quello che è stato, credo che di Berlusconi sia rimasto in tutti coloro che lo hanno apprezzato un grande, grandissimo rispetto. Grazie Silvio per il ricordo che ci hai lasciato.

membro del Governo, Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, con un grande impegno per cercare di rinnovare il nostro Paese. Penso alla legge obiettivo; penso alle tante scelte, come la prima di digitalizzare l'Italia per renderla più competitiva; penso alla scelta di far sì che le nostre ambasciate fossero luogo di promozione per le nostre imprese nel mondo. La forte vicinanza agli Stati Uniti, da chiunque fossero governati. Ricordo il suo discorso al Congresso. Divenne un fatto memorabile, invitato dal Presidente degli Stati Uniti a parlare. E lui ricordò l'impegno dei giovani americani che combatterono per la libertà dell'Italia

di Tblisi da parte dell'armata della Federazione Russa. E anche il dispiacere per un atteggiamento, che non condivideva più, di quello che lui considerava un amico, qual era Putin. Diceva sempre: "è un uomo che è cambiato". Al Parlamento europeo votò contro l'invasione dell'Ucraina, insieme a tutti quanti noi, a dimostrazione che prevalevano i valori dell'Europa e della libertà, rispetto anche a quella che era stata l'amicizia con un *leader* politico. Per lui non contavano i colori politici, contavano soprattutto i rapporti personali. Certamente difendeva le sue idee in politica estera: l'europeismo, l'atlantismo. Era sempre pronto a confrontarsi con chiunque, pur di tutelare l'interesse nazionale, rispettando sempre e comunque le persone. Anche come uomo di Governo, ha sempre voluto confrontarsi con le opposizioni. Ricordo che una volta - ero Capogruppo al Parlamento europeo - c'era un'autorizzazione a procedere nei confronti di Massimo D'Alema. Lui ci telefonò e disse: "votate come se fossi io al posto di Massimo D'Alema". A dimostrazione che era garantista non per la sua persona, ma per chiunque dovesse affrontare dei giudizi. Così come scelse di partecipare all'ultimo Governo di unità nazionale nell'interesse superiore dell'Italia, sia pure con perplessità. Anteponeva sempre, da uomo di Governo, da Ministro degli esteri e da *leader* di partito, l'interesse nazionale a qualsiasi altra cosa. Decise anche di partecipare all'ultimo Governo prima dell'attuale, quello guidato da Mario Draghi, in compagnia di forze con le quali non condivideva le scelte valoriali e ideali; ma c'era l'interesse dell'Italia. Così come ricordo - e mi spiace che non ci siano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle - che anche nei confronti di Conte Presidente del Consiglio ebbe sempre e comunque un atteggiamento rispettoso, perché, pur non essendo il il presidente Conte in sintonia con le sue posizioni, però rispettava sempre l'istituzione, cosa che non è comune di questi tempi, il rispetto ci deve essere sempre, anche dell'avversario politico. Qui non si tratta di combattere le persone *(Applausi)*, ma si tratta di combattere semmai le idee, rispettando sempre e comunque le persone, a maggior ragione quando queste persone non ci sono più. Rendo omaggio al Presidente del Consiglio più longevo della storia della Repubblica. Rendo omaggio al Ministro degli affari esteri. Rendo omaggio al *leader* politico che ha fatto del rispetto degli altri il centro della sua attività personale e che ha fatto della difesa dei suoi valori, primo fra tutti la libertà, il centro della sua attività politica. *(Applausi)*. Non mi resta che rivolgere un pensiero ai suoi familiari, a Marta, Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora, Luigi e ai suoi nipotini e chiedervi qualche secondo di raccoglimento

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 4 luglio. Restano confermati gli argomenti già stabiliti per la settimana corrente: seguito della discussione del disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e discussione del disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza. Per il disegni di legge costituzionale la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di ampliare i tempi del contingentamento, su mia proposta, attribuendo ulteriori due ore complessive ai Gruppi di opposizione che l'hanno richiesto. Per il disegno di legge sulla cybersicurezza si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per un totale di tre ore e trenta minuti escluse le dichiarazioni di voto. Il calendario della prossima settimana, che sarà con eventuali sedute senza orario di chiusura, a partire da martedì 18, alle ore 11,30, prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi questa settimana, nonché il decreto-legge coesione. Alle 15,30 di martedì 18 giugno avranno luogo le dichiarazioni di voto finali, con trasmissione diretta televisiva del disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. settimana dal 25 al 27 giugno sarà discusso, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, il decreto-legge in materia di rappresentanze sindacali militari attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Nella mattinata dello stesso mercoledì 26 la presidente Meloni consegnerà al Senato il testo delle comunicazioni rese poco prima alla Camera dei deputati. Nella settimana dal 2 al 4 luglio sarà discusso il decreto-legge in materia di agricoltura e imprese di interesse strategico. Nelle sedute di giovedì 27 giugno e di giovedì 4 luglio,

è convocato il Parlamento in seduta comune, alla Camera, per la quinta votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli

Presidente, confidavo nella sua grande saggezza. PRESIDENTE. Io confidavo che lei ci avesse ripensato. Come abbiamo sottolineato nella Conferenza dei Capigruppo, il Gruppo Partito Democratico, ma immagino anche gli altri Gruppi di opposizione, ha chiesto ripetutamente l'inversione dell'impianto che la maggioranza ci sta proponendo perché, come avevamo già sottolineato nella giornata di ieri, il decreto-legge sulla cybersicurezza è stato rappresentato rappresentato a metà. Come è noto è stato espunto di altri pezzi che arrivano attraverso un altro provvedimento e già di suo è difficilmente comprensibile. Se poi il nostro Governo, ritiene di potersi presentare al tavolo dei grandi della terra con un decreto-legge così pasticciato e, tra l'altro, votato in fretta e furia in Commissione affari costituzionali

prendiamo atto del tempo extra che è stato dato alle opposizioni, ma riteniamo che non sia sufficiente né adeguato. Sappiamo inoltre della sua disponibilità - gliene abbiamo dato atto - per eventuali allungamenti, ma il tema non è allungare allungare di un quarto d'ora o di mezz'ora la disponibilità al confronto, che però è unilaterale. Il tema vero è che manca la maggioranza: noi parliamo, facciamo richieste, poniamo temi, ma la maggioranza non risponde e non abbiamo capito se non lo fa perché deve obbedire al Governo o se questo è l'unico atteggiamento possibile che la maggioranza ha deciso di avere sulla riforma della nostra Costituzione. Pertanto insistiamo, insisteremo ancora e continueremo a farlo, ovviamente lo facciamo ora in questo snodo della definizione del nuovo calendario. Ribadiamo che un'ora, due ore o tre ore in più

che un Presidente del Consiglio (perché per voi c'è solo un'idea di Presidenza del Consiglio) debba avere il potere di scegliere e sciogliere il Parlamento; noi continuiamo a essere legati all'idea che sia il Parlamento a scegliere il Governo e il Presidente della Repubblica a sciogliere eventualmente il Parlamento. Siamo distanti, continuiamo a chiedervi il ritiro del provvedimento, lo faremo con tutti gli strumenti democratici a disposizione e ovviamente questo passa anche attraverso

Signor Presidente, esprimo da parte nostra il sostegno alla proposta del presidente Boccia. Ricordo, peraltro, che

Presidente, intervengo a nome del mio Gruppo per appoggiare la proposta avanzata dal presidente Boccia e per associarmi anche alle valutazioni, che sono oggettivamente condivisibili, portate sia del presidente Boccia, sia dal presidente Patuanelli innanzitutto sul tema dell'urgenza di questo disegno di legge sulla *cybersecurity*, che sicuramente è un provvedimento importante e urgente, visto che il Governo ci ha spiegato e ha condiviso l'esigenza di approvarlo prima del G7, ma non capiamo come mai, se non capiamo come mai, se è così urgente, non ce ne stiamo occupando e stiamo invece votando un provvedimento come la riforma costituzionale che non solo non ha scadenza, ma addirittura deve attraversare almeno quattro letture a distanza di tre mesi l'una dall'altra, quindi non sarà un giorno in più o un giorno in meno a fare la differenza. Se è urgente la *cybersecurity*,

che oggi ci sono state concesse un paio d'ore in più di discussione, che a me non sembrano congrue, perché stiamo discutendo un provvedimento importante, lo dico ancora una volta da parte di un Gruppo che non ha una chiusura pregiudiziale, ma ci sono ancora dei nodi di questa riforma che vanno discussi e sarebbe bene che approfittassimo di questo tempo per provare a fare qualche modifica migliorativa sulle questioni di merito che ancora, anche a giudizio degli studiosi, sono sul tappeto.

argomento: qui si discute sulle modalità di elezione ed è, in realtà, lo stesso argomento dell'articolo 5, cioè la questione dell'elezione per trascinamento di entrambi i rami

trascina la stessa composizione del Parlamento. Vorrei tornare su un argomento che è stato più volte trattato, cioè il fatto che, nella situazione che stiamo vivendo da anni, come da ultimo ci confermano le percentuali di votanti alle elezioni europee, si sarebbe aspettati un dibattito dedicato in Aula, una grande discussione, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le forze politiche

Ieri sera, con sorpresa, in un *talk show* televisivo, un esponente della maggioranza, su questo punto su cui si era animata molto la discussione, ha affermato,

questa è la riprova che si vuole una democrazia di oligarchi, di pochi, mentre la cifra che si vuole caratterizzante di questa maggioranza, in particolare del partito di maggioranza relativa, è quella del popolo, evocato un giorno sì e l'altro pure,

cioè il problema della partecipazione dei cittadini, che è crollata e che è una questione che dovrebbe coinvolgerci tutti. Quelli che non votano, tra l'altro, sono esattamente i ceti più popolari, chi è più in difficoltà. Questo principio si preoccupa o non si preoccupa di ciò? Qui c'è un tema, quindi. È su questo presupposto che la questione della rappresentanza diventa cruciale ed è uno dei punti della riforma dell'articolo di cui stiamo discutendo. Su questo discorso, nel momento in cui la partecipazione è crollata e vi è un grande astensionismo di cui nessuno si fa carico, si innesta un meccanismo che spezza verticalmente il concetto di rappresentanza, che già è stato innescato. Il dibattito di questi ultimi anni sui sistemi a tendenza maggioritaria si colloca esattamente nel punto di equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Ora, con questa vostra riforma, sganciate completamente il concetto di rappresentanza dal modello di democrazia: questo è il punto. Per questo diciamo che voi

vuoto: è la crisi verticale delle democrazie, di qualsiasi democrazia. Questo è il punto fondamentale su cui noi vorremmo che ci deste delle risposte. Quando diciamo che volete riscrivere la Costituzione, intendiamo che volete riscrivere l'idea di democrazia; una democrazia che, a usare termini generosi, è elitaria ed escludente e sicuramente non ha niente a che vedere con il popolo.

Questo fa parte di un andazzo, nel senso che non è la prima volta in questi anni che si sposta la soglia di attenzione tutta sul tema della stabilità di Governo, che pure è reale, esiste e nessuno lo nega. Si mortifica radicalmente e completamente però quello che perlomeno dovrebbe essere l'altro corno della discussione. Stabilità e rappresentanza dovrebbero perlomeno meritare una trattazione comune. comune. Invece, da molti anni a questa parte, siamo arrivati al punto finale di questo percorso: il tema della stabilità è diventato una sorta di pensiero unico, di mantra attorno al quale è stata definita una narrazione: il Paese non funziona perché ci sono troppi Governi e perché c'è poca stabilità. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Migliaia, nel corso di questi anni. Abbiamo sentito però molto di meno l'altra frase che invece meriterebbe perlomeno un'eguale attenzione: il Paese non funziona perché le forze politiche sono sempre meno rappresentative e la popolazione italiana va sempre meno a votare. Io penso - lo sto dicendo e mi sto sgolando su questo punto da molte settimane a questa parte - che avremmo dovuto centrare tutta l'attenzione su questo punto, ossia sul tema grande, gigantesco della rappresentatività. Avremmo dovuto farlo anche mettendo in discussione alcune idee che sono state presentate come dogmi nel corso di questi decenni e che però, francamente, di dogma non hanno nulla, o meglio vengono presentate come tali, ma sono invece suscettibili di critiche molto semplici. Ad esempio, ritengo che contenere nelle stesse leggi elettorali due princìpi totalmente contraddittori - o, meglio, due princìpi che messi insieme mortificano la rappresentanza, cioè il premio di maggioranza e gli sbarramenti - sia una cosa che, anch'essa, non esiste da nessuna parte. O c'è il premio di maggioranza, quindi non c'è lo sbarramento, oppure c'è lo sbarramento, quindi, come in Germania, non c'è il premio di maggioranza. Tenere insieme queste due cose è stata una delle caratteristiche del sistema politico italiano di questi ultimi trent'anni ed è stato esattamente il segno di quella distorsione maggioritaria sulla quale avremmo dovuto definire e costruire oggi una vera presa di posizione (o, meglio, avremmo dovuto costruire un ragionamento). È possibile che in questo Paese non si possa fare un bilancio su ciò? Faccio riferimento al maggioritario o alle leggi proporzionali con distorsioni maggioritarie, poiché quelle con cui votiamo oggi sono soltanto apparentemente leggi proporzionali, mentre sono in realtà profondamente maggioritarie nell'impianto distorsivo che presentano. Il maggioritario introdotto in Italia nel 1993 ha migliorato la tenuta sociale di questa democrazia oppure no? Io penso che questa sia una domanda rispetto alla quale ognuno di noi dovrebbe riflettere molto seriamente, cercando di fare un passo indietro anche rispetto alla propria posizione politico-culturale di fondo. Io, che sono sempre stato un proporzionalista, mi sono molto interrogato nel corso di questi anni se per esempio alcune sperimentazioni che sono state fatte, una per tutte le primarie, che non hanno niente a che fare con la storia dei sistemi proporzionali, non potessero effettivamente portare, almeno in alcune fasi, degli elementi di giovamento. Penso che una tale riflessione andrebbe fatta e in qualche modo articolata. La cosa che trovo davvero incredibile è che si continui con questo elemento dogmatico. Queste leggi elettorali, questi premi di maggioranza abnormi, in altri anni, Presidente, sono state chiamate leggi-truffa, perché un tempo, quando esisteva nel nostro Paese la democrazia dei partiti, le distorsioni maggioritarie e i premi di maggioranza venivano chiamati così e non in un altro modo. Ebbene questi meccanismi, l'attribuzione cioè di un numero di seggi, che molto spesso è diventato quasi equivalente al peso... ...dei partiti nella società, io credo avrebbe meritato un'indagine seria e invece andiamo avanti come l'orchestra che suonava mentre il ghiacciaio si avvicinava.

provare un sentimento di orrore di fronte a un tale stravolgimento della Carta fondamentale. La Costituzione è stata concepita come un'opera di ingegneria giuridica di diritto costituzionale ed è stata costruita con una genialità che ha consentito ai Padri costituenti di stabilire una serie di equilibri, di pesi e di contrappesi che hanno consentito di proteggere i diritti dei cittadini e di garantire la democrazia, nonché di proteggere gli italiani da qualsiasi pericolo di una deriva autoritaria. Questa riforma è l'antitesi del diritto. Sembra quasi più un esercizio dilettantistico basato su una confusione di princìpi e, piuttosto che sulla conoscenza delle norme di diritto costituzionale, su una sorta di diritto per sentito dire, il diritto di pancia, che vuole consentire di stravolgere i princìpi cardine della democrazia. Infatti, il

nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, ed è considerato da tutti gli Stati europei come un principio fondamentale e fondante? Come si può conciliare questo squilibrio costituzionale con lo Stato di diritto e l'esigenza di bilanciamento dei poteri, senza i quali non si può parlare di democrazia? A questa domanda ci dovete rispondere, perché la stiamo ponendo da tempo, sia in sede di Commissione sia qui in Aula, ma non abbiamo ricevuto risposta e sapete perché non c'è risposta? Perché non è possibile rispondere a questa domanda,

voi che dovreste avere una cultura giuridica, come fate a concepire una norma che tutt'al più può essere inserita all'interno di una legge elettorale? È una distorsione democratica: voi state costituzionalizzando costituzionalizzando la possibilità di un governo di minoranza, che si basa su una duplice distorsione democratica, perché il *Premier* che farà riferimento a una forza politica minoritaria avrà l'appoggio di altre forze politiche con le quali si farà un accordo di massima, anche se i programmi sono divergenti, e poi ci sarà il premio di maggioranza. E questo lo considerate un principio da inserire nella Carta fondamentale, nella nostra Costituzione? Non credo che ci sia la possibilità, da giuristi, di accettare una cosa del genere. Ve lo dimostra un fatto: su una rivista di diritto

vorrei dire che sono contraria su tutti gli emendamenti, perché l'articolo 6 prevede che il premio di maggioranza, che viene assegnato al Senato su base nazionale e non regionale, superi quell'asimmetria che c'è sempre stata fra Camera e Senato e che ha dato luogo in passato a complessi problemi di carattere applicativo. Vorrei anche cogliere l'occasione per fare eco a quello che diceva stamattina, di fronte alle vostre ripetute domande, il senatore Lisei intorno alla legge elettorale. Continuate a chiedere perché non non abbiamo scritto prima la legge elettorale e dite continuamente che non avete avuto delle risposte. Non è così, perché sia in Commissione, sia in Aula, nelle repliche ho detto che avrei costruito la legge elettorale nel passaggio dal Senato alla Camera, quando ci fosse stata quantomeno un'ossatura della riforma. mi sembrava infatti di ingessare la riforma costituzionale con paletti troppo rigidi rispetto ad un dialogo che mi immaginavo ci fosse realmente. E qua davvero mi stupisce il richiamo continuo che si fa in quest'Aula, dicendo che tanto la maggioranza quanto il Governo sono silenziosi. da un lato protestate perché non c'è la legge elettorale, dall'altro continuate a dire che questa legge porterebbe una sorta di elezione a strascico. Come fate ad affermare questo, se non c'è una legge elettorale? Come fate a dire che c'è una legge a strascico, quando dell'elezione non sapete o dite di non sapere? Fate un'affermazione assolutamente aporetica, di fronte al fatto che è scritto soltanto che ci sarà. Forse chiedete risposte, però poi non sapete ascoltare. che il senatore Lisei ha spiegato il perché della mancata riforma elettorale, è intervenuto il senatore Giorgis, che io stimo profondamente. Ma non ho capito perché si fanno delle domande, si ottengono delle risposte e la controrisposta è di nuovo la domanda. Allora, non ci siamo: non è certamente non è certamente un ragionamento hegeliano (tesi, antitesi e sintesi: di solito, si fa così).

di riforma o con che tipo di ragionamento stiamo discutendo, perché c'è un silenzio quasi assordante. Ma io posso rispondere su

si fa tutta una lista di numeri che nulla hanno a che fare con il contenuto di questa riforma? Io avrei voluto discutere su una proposta alternativa che non c'è stata, non sui numeri, non su questo. *(Applausi)*. In effetti, il senatore De Cristofaro,

da parte di chicchessia per una legge che non ha e non prospetta alcuna deriva autoritaria, nessuna lacerazione della Carta costituzionale.

la piattaforma per qualsiasi cosa e non si consulta per la scelta di chi dovrà venire a governarci? Mi stupisce! Avete detto che non ho mai parlato: vorrei parlare. Il MoVimento 5 Stelle si dimentica forse, quando parla di svilimento del Parlamento, che che una delle sue proposte tipo era il *referendum* propositivo che andava ad eliminare la funzione del Parlamento e la democrazia rappresentativa? *(Commenti)*. Ci siamo dimenticati

elimina totalmente o quasi il ruolo proprio del Parlamento, quel ruolo che dite di difendere a parole *(Applausi)*, ma che di fatto non sostenete. Ho sempre dimostrato una grande disponibilità, ma sul merito, non sui numeri 1.000 emendamenti ostruzionistici, senza alcuna proposta alternativa. Noi abbiamo mantenuto tutte le prerogative del Capo dello Stato. Per quanto che vagheggia un cancellierato alla tedesca, tutti sanno bene che il Presidente della Repubblica tedesco ha zero poteri rispetto al Parlamento. Allora bisogna dire la verità ai cittadini che ci ascoltano, perché solo su di essa possiamo costruire insieme, come sarebbe dovuto essere e ho tentato di fare. Nel nostro programma c'era infatti il semipresidenzialismo:

tipo di ira, come ho visto che può accadere. Abbiamo degli emendamenti da votare, interverremo su quelli, quindi non voglio crearle problemi.

la caratteristica di un intervento di ripristino della verità non politica, ma dei fatti, che è stata maltrattata nell'intervento della Ministra, come mai ho visto fare in quest'Aula in tanti anni.

Presidente, quando il Governo interviene con un intervento politicamente molto pesante, le opposizioni non possono che interloquire, non è che possono star lì lì ad ascoltare. Peraltro, la Ministra ha detto delle cose importanti e, se non ci viene data la parola, come di solito accade, per commentare l'opinione della Ministra, utilizzeremo i minuti che generosamente sono stati *octroyé* dal presidente La Russa al mio Gruppo per rispondere al Governo. [DE

perché fa parte delle prerogative di un senatore) che, se vengo citato dal Governo, devo essere citato sulla base delle cose che dico e non sulla base delle cose che al Governo fa comodo che vengano dette. *(Applausi)*. Dico pertanto alla ministra Alberti mi dispiace, ma evidentemente non mi ha ascoltato in tutte queste settimane, non mi ha ascoltato in Commissione: che le devo dire? Forse è distratta quando parlano le forze politiche più piccole, magari si vada a guardare i dati elettorali, così si accorge che non sono nemmeno così piccole, quindi la invito ad ascoltare meglio. In ogni caso, attribuire alla mia forza politica di aver presentato esclusivamente emendamenti ostruzionistici è una inaccettabile forzatura della realtà. Ho sempre rivendicato in quest'Aula di aver presentato molti emendamenti ostruzionistici, perché li ritengo un diritto, quando si difende la Costituzione, come in questo caso.

secondo la quale nel modello tedesco in Germania i poteri del Presidente della Repubblica sarebbero - secondo lei - limitati, poi le spiego perché probabilmente non avete capito come funziona il modello tedesco

la ministra Casellati, che ha parlato di tutto, non solo dell'articolo 6, è partita da quello e ha fatto una serie di valutazioni anche di merito sul comportamento dei Gruppi parlamentari di opposizione che, se lei mi permette, non è compito della Ministra, al limite sarebbe compito del Presidente se ritenesse di dire alcune cose, ma non lo farebbe mai il Presidente. Noi pensiamo, presidente Centinaio, che forse in questo momento consentire ai Gruppi di opposizione di intervenire per cinque minuti a Gruppo per ripristinare la verità sull'articolo 6 e anche per rispondere alla Ministra possa migliorare il clima già surriscaldato di quest'Aula. Le sto facendo una proposta da pompiere, presidente Centinaio, e non da incendiario. Signor Presidente, mi dispiace aver perso gran parte dell'intervento della ministra Casellati e non ho capito quindi a che titolo interveniva e quindi cosa provoca qui all'interno dell'Aula. PRESIDENTE. Stava dando il parere sugli Non si è limitata, però, a dare il parere sugli emendamenti, ma ha espresso opinioni politiche anche rispetto alla democrazia interna dei Gruppi presenti in Aula anche rispetto alle proposte emendative avanzate dai Gruppi di opposizione. Mi sembra che si sia spinta molto oltre quello che è il ruolo che le competerebbe, ossia di esprimere opinioni di merito e pareri sugli emendamenti. Visto che ci siamo entrati, entrati, non consento a nessuno di mettere in discussione il concetto di democrazia del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. Questo anche perché - voglio rinfrescare la memoria a tutti i colleghi e le colleghe presenti non significa semplicemente andare a votare una volta all'anno per una persona, ma democrazia è partecipazione, è consentire alle persone di partecipare ai processi decisionali dall'inizio fino alla fine *(Applausi)*, cosa che voi avete respinto, bistrattando le leggi di iniziativa popolare che qui in quest'Aula avete affossato, per esempio quella rispetto alla modifica del Titolo V della Costituzione, anche se poi però andate in giro a dire che non l'avete voluta voi la modifica del Titolo V nel 2001, ma l'ha fatto qualcun altro e quando avete avuto la possibilità di cambiarlo, ovviamente l'avete gettata *(Applausi)*. Noi abbiamo proposto anche il rafforzamento del *referendum* abrogativo e anche del *referendum* propositivo, che non significa bypassare il Parlamento, perché bypassare il Parlamento, anzi abolirlo è quello che fate voi, concentrando il potere di vita o di morte nelle mani di una sola persona eletta una volta ogni cinque anni per due mandati, eventualmente due mandati e mezzo. *(Applausi)*. Dopodiché, questa potrebbe anche cambiarsi le regole in gioco e rendere il suo un regno potenzialmente infinito e perpetuo, come succede in Russia, come succede in Ungheria, come succede in Turchia. Non andate, Non andate, allora, a cacciarvi in questi impicci, a parlare di democrazia rispetto al mio Gruppo in particolare, perché mi sembra che di problemi rispetto al concetto di democrazia ne abbiate voi. Il problema più grande che ha questo Paese è che le vostre menzogne stanno coprendo la realtà di questo pateracchio che avete avuto il coraggio di scrivere e di presentare addirittura in Aula, che tutti i costituzionalisti vi hanno detto che è un abominio che non sta né in cielo né in terra, ma che vi ostinate a voler far votare. Tanto il popolo italiano ve lo boccerà.

che la norma per la quale se il Governo interviene riapre la discussione si applica, come dice la parola, alla discussione generale. Questo è, basta leggere il Regolamento. *(Commenti).* Lasciatemi parlare, visto che non avete lasciato parlare il Ministro, sommergendola di ululati e di muggiti. Eravamo in una fase molto semplice: erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 6,

Ma la regola non è che, se non siete d'accordo voi, voi potete fare tutto quel che volete e, quando non siamo d'accordo noi, dobbiamo stare zitti. Questa è una regola che abbiamo visto tante volte aleggiare in molti interventi. *(Applausi)*. Noi stiamo facendo cose molto simili a cose già fatte da voi. Però, se le facciamo noi, è sbagliato; quando le facevate voi, erano giuste, non c'era alcuna discussione, nessuno metteva in dubbio che gli interventi sull'ordine dei lavori, i richiami al regolamento nel corso di una discussione con i tempi contingentati facessero parte del tempo contingentato, il sistema del canguro, non lo ha mai messo in discussione nessuno. Adesso il canguro non si può fare e i tempi contingentati dovrebbero interrompersi. Le regole in democrazia

un testo alternativo lei lo ha. È a firma del senatore Renzi e sta dentro il fascicolo, nel senso che questa parte dell'opposizione ha presentato un disegno di legge costituzionale. Quindi, non è vero che non c'è stata una proposta alternativa. In secondo

che quello che sta succedendo qui è normale amministrazione in una democrazia parlamentare. Non c'è niente di scandaloso in questo, nel senso che le opposizioni fanno l'opposizione, con tutti gli strumenti che hanno, anche Le assicuro che, in Governi precedenti, chi era seduto al suo posto riceveva il lancio fisico del Regolamento del Senato. Io ne ho schivati vari, spostandomi con una certa rapidità che poi, con l'età, ho perso. Quindi, quello che sta succedendo qui, in una discussione così importante, è normale. Io vorrei anche che il Ministro riassumesse la *gravitas* necessaria per ricoprire il ruolo.

dopo la prima lettura del Senato e che, quindi, noi non sappiamo. Il problema, signor Ministro, è proprio che noi non sappiamo e che lei ci chiede di votare nel momento in cui noi non sappiamo. Probabilmente, se sapessimo, avremmo anche la possibilità di decidere. Come si dice: conoscere per deliberare. Lei, però, viene in quest'Aula con un testo criptico, che non spiega che cosa farete. Io le vorrei chiedere, per esempio: facciamo il ballottaggio, sì o no? Mi basterebbe anche questo. Abbiamo la garanzia che il Presidente del Consiglio sia eletto dalla maggioranza più uno degli elettori o vi è la possibilità che il Presidente del Consiglio sia espressione di una minoranza degli elettori e goda della maggioranza sulla base di un meccanismo di premialità che sarebbe a questo punto incostituzionale? Mi accontenterei anche solo di questo. Come vede, mi accontento di poco, ma purtroppo non lo so. Allora, nonostante tutta l'apertura del mondo ed il desiderio di contribuire alla riforma costituzionale, di cui io credo che noi abbiamo molto bisogno, le dico che, su questa base, è difficile. Quindi, non se ne abbia a male se facciamo opposizione: è normale. Lei non è la prima a passarci e, avendo ricoperto la carica di Presidente di questa Camera, sa bene come funzionano le cose. Io credo che siamo nel normale svolgimento fisiologico della nostra democrazia. Se ci aiutate, facendoci capire meglio, vedrà

di sciogliere il Parlamento, che può tenerlo sotto ricatto, che non può essere sfiduciato senza che si sciolgano le Camere. Lei ci dice che non è un'elezione a strascico, ma la regola del *simul simul* che altro significato può avere? Fatta questa premessa, parliamo anche in questo caso di un articolo soppressivo e su tutti gli articoli soppressivi noi votiamo convintamente a favore, perché siamo dell'idea che questa questa riforma truffa i cittadini e viene presentata come un *aliud pro alio*. State vendendo qualcosa che non è la realtà di questa riforma. State continuando a illudere i cittadini che possano scegliere loro stessi quella stessa figura istituzionale che sono abituati a a conoscere, ma non è così. State nascondendo tutti gli altri punti essenziali della riforma, come quello del premio di maggioranza che vorreste inserire nella Costituzione. Se volete inserire in Costituzione una stortura democratica come questa, almeno fatela bene. Avete messo un premio di maggioranza senza dire quando viene assegnato. Quindi cosa vuol dire? Può essere assegnato se si raggiunge il 25 per cento, oppure Penso che, se inserite il premio di maggioranza in una legge elettorale, occorra chiarire anche quando questo può essere assegnato. Se lo inserite nella Costituzione - e state commettendo un errore dal punto di vista giuridico -, dovete chiarire anche in quando può essere assegnato. Altrimenti, costituzionalmente parlando, rendereste legittima qualsiasi legge elettorale preveda un premio di maggioranza, salvo un nuovo intervento della Corte costituzionale, a questo punto, confermare che bisogna garantire almeno un 40 per cento, oppure, visto che c'è stata una riforma, non riusciamo a prevedere in questo caso che cosa si potrà dire. Abbiate il coraggio di dirlo. Fate una riforma, inserite un premio di maggioranza, dite quando e dite anche quanto: quanto può essere costituzionalmente accettabile un premio. È inutile che usate parole come «rappresentatività»; cancellate quella parola, perché è un'ipocrisia, è l'ennesimo inganno dei cittadini. cittadini. Alla fine, i cittadini non sceglieranno niente, perché ci saranno le manovre preventive di palazzo, che stabiliranno a tavolino quale coalizione si farà, con un'accozzaglia di programmi, per avere un premio di maggioranza e creare un governo di minoranza che avrà pieni poteri e potrà sciogliere il Parlamento quando vuole. siamo rimasti molto preoccupati dall'intervento della ministra Casellati. Siamo molto, molto preoccupati e cercherò di spiegare perché. Siamo preoccupati per quello che la Ministra si è rifiutata di dire e preoccupati per quello che la Ministra ha detto. La Ministra si è rifiutata, in un intervento molto articolato ed ampio, di rispondere alla domanda più importante che le è stata fatta durante tutta questa discussione; una domanda alla quale si poteva rispondere - adesso lo spiegherò - con dieci o con sette parole.

eleggere direttamente un Presidente del Consiglio con molti poteri a colpi di minoranza. Lei a questa domanda poteva rispondere con dieci parole dicendo: noi non vogliamo eleggere un *Premier* a colpi di minoranza. Oppure poteva rispondere con sette parole: noi non vogliamo una capocrazia Ha scelto di non dare alcuna risposta a questa nostra domanda e questa omissione è molto sospetta, molto grave e dice sulla natura delle vostre intenzioni riformatrici più di quanto si immagini. Noi siamo costretti, ancora una volta, a sottolineare questa fuga dai quesiti che l'opposizione pone e la fuga dai quesiti che l'opposizione pone non è mai una buona cosa per la qualità del dibattito parlamentare. Quello che lei ha detto ci preoccupa ancora di più. Noi dovremmo, pur nella diversità delle idee, essere d'accordo sul significato delle parole. Lei ci ha spiegato che non è vero che il Parlamento viene eletto a strascico, ma noi, di fronte a questa affermazione, sobbalziamo perché o ci sono stati consegnati dei testi falsi oppure noi leggiamo all'articolo 5 che la legge disciplina il sistema per le elezioni delle Camere del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. quello che succede alla composizione del Parlamento è un fatto automatico determinato dall'elezione del Presidente del Consiglio, significa che l'elezione del Parlamento non è autonoma, ma è il prodotto di un automatismo e quindi significa che è a strascico. *(Applausi)*. Ci dica nel prossimo intervento, quando interverrà sui pareri all'articolo 7 parlando di tutti gli articoli della riforma, che cosa intende lei per "a strascico". Noi in questa opera di chiarificazione delle nostre posizioni le diciamo che si dice Parlamento eletto a strascico tutte le volte che l'elezione del Parlamento non è autonoma, ma è determinata da un'altra elezione. Voi avete scritto un articolo che dice esattamente questo, quindi, almeno sui fatti, dovremmo metterci d'accordo. *(Applausi)*. Seconda cosa che cerco di spiegarle con la massima calma: per tutta la politologia contemporanea, se si paragona la forma di governo di un Paese a un edificio, tutti i politologi dicono che le fondamenta di quell'edificio sono date dalla legge elettorale, il primo piano dal sistema politico e il secondo piano dalle norme costituzionali. senza far torto a tanti anni di scienza, non può permettersi di dirci che la legge elettorale è cosa diversa dall'ossatura della forma di governo di un Paese. La legge elettorale è parte essenziale della forma di governo di un Paese. Lei sta trattando come un orpello e un ornamento quello che è un elemento fondamentale dell'architettura della nostra democrazia, ed è per questo che il rifiuto di parlare di legge elettorale è un'offesa a questo Parlamento. Inoltre, nonostante tante nostre avvertenze in questo senso, si continua con il maltrattamento dei sistemi costituzionali degli altri Paesi perché fare la caricatura dei sistemi costituzionali degli altri Paesi io credo che porti male, prima di tutto, e poi non è nemmeno rispettoso sul piano delle relazioni internazionali. Inoltre, signora Ministra, mi è parso anche sfortunato, per il momento in cui avviene, l'accenno che ha fatto, al fatto che il semipresidenzialismo francese annullerebbe l'autonomia del Parlamento rispetto al Presidente della Repubblica, perché leggendo i giornali di questi giorni tutto il mondo pensa che la Francia... *(Il Tutto il mondo si aspetta che la Francia il 14 luglio, dopo che si sarà tenuto il secondo turno delle legislative, avrà un Parlamento con una maggioranza di colore opposto a quella del Presidente della Repubblica, quindi ha detto una cosa non solo falsa, ma che sarà prestissimo dimostrata falsa. *(Applausi)*. il Presidente della Repubblica tedesca abbia zero poteri. Signora Ministra, le Costituzioni non sono testi segreti a cui solo lei ha accesso, si trovano su Internet. All'articolo 63 della Costituzione tedesca, è scritto che il cancelliere è eletto dal Bundestag su proposta del Presidente federale. Al secondo comma di quell'articolo è scritto che se il Cancelliere non ha la maggioranza assoluta, la decisione insindacabile se far partire il suo Governo o sciogliere le Camere è del Presidente della Repubblica, e questo potere è paragonato dai costituzionalisti a una bomba atomica. L'articolo 68 dice che se il *Premier* propone lo scioglimento, il Presidente della Repubblica... Grazie senatore, le ho già dato un minuto in più. *(Commenti)*. Tanto discende il tempo, io non ho problemi. Per me potete parlare anche due ore; poi, quando non ne avete più, non ne avete più. Un minuto, va bene. L'articolo 68, che regola la procedura di scioglimento anticipato delle Camere, dice che in Germania questa può essere proposta dal Cancelliere, ma il Presidente della Repubblica può rifiutare la proposta del Cancelliere, mentre voi ci proponete un sistema in cui il *Premier* propone lo scioglimento e il Presidente della Repubblica ha solo il potere di ratificare la volontà del Presidente del Consiglio. Quindi che in Germania il Presidente della Repubblica abbia zero poteri non è una cosa che si può discutere: è una palese panzana e sarebbe meglio non dire le panzane.

che in politica si può far finta di nulla, ma poi i problemi riemergono alla prima curva. La discussione a cui stiamo cercando cercando di dare corpo con diverse voci questo pomeriggio si sarebbe tranquillamente potuta evitare e voi l'avreste potuta risolvere se aveste avuto la lungimiranza politica di accogliere un ordine del giorno che noi avevamo rappresentato all'inizio di questa discussione.

arrivare al voto finale della riforma costituzionale in assenza di una legge elettorale approvata che sia coerente con il contenuto della riforma costituzionale. Noi abbiamo soltanto proposto questo minimo sindacale, che avrebbe consentito a questa Camera un'attività di esame quantomeno sotto la copertura del vincolo di un impegno politico. Questo non è avvenuto, ma si è inteso procedere a fari spenti nella notte, immaginando di farsi dare un *affidavit* da parte della maggioranza, che quindi ritiene di dare al Governo e alla sua *Premier* una sorta di cambiale, che naturalmente, signora Ministra, è a scadenza, è a scadenza, in connessione con alcuni impegni che vi siete assunti sotto altri versanti. Penso all'autonomia differenziata, penso alla riforma della giustizia, dentro un concatenamento che prima o poi arriverà Ma la questione rimanda anche a una concezione un po' più strutturata. Voi ci state proponendo di cambiare costituzionalmente la natura della nostra rappresentanza politico-parlamentare. Questo tema significa voler trasferire sul versante delle geometrie istituzionali questioni che attengono ai rapporti politici. La La formazione delle maggioranze e delle alleanze tra forze politiche non dovrebbe essere la conseguenza di una camicia di forza stabilita da una regola costituzionale, ma dovrebbe essere la libera interpretazione scelta da parte delle forze politiche, che, partendo da una condivisione sui contenuti, sui programmi e sugli obiettivi, arrivano a stipulare delle alleanze sulle quali chiedere il consenso e sulle quali, se si ritiene, ragionare in termini di possibile premio di maggioranza. Voi non state facendo così. Voi state facendo l'opposto, state costruendo una camicia di forza dentro la quale le forze politiche attuali e di domani saranno costrette ad infilarsi, prescindendo dagli elementi di merito. Il risultato è sotto gli occhi di tutti quotidianamente. Pensate a un tema così dirimente, qualificante e preoccupante come il tema della guerra e della politica estera. Oggi i due schieramenti, che dovrebbero nascere in nome del rosso e del nero, del bipolarismo forzato, della riduzione a due, su questi temi, a destra come a sinistra, sono spaccati come una mela al loro interno. Questa è la dimostrazione plastica che quando si pretende di trasferire i processi politici alle geometrie istituzionali, ad un certo punto, il sistema non regge più. Ciò accade perché voi state semplicemente espungendo l'elemento fondamentale della politica, che è quello della gestione della complessità, pensando che essa sia la *reductio ad unum* o al massimo a due.

l'ordine dello Stato con l'intima libertà del cittadino, che esprime il massimo del suo diritto di cittadinanza nel momento in cui va a votare.

con altri Paesi europei e con altri sistemi istituzionali che esistono da altre parti d'Europa) di non citare a sproposito i modelli istituzionali degli altri Paesi. Il senatore Parrini ha citato gli citato gli articoli della Costituzione che in Germania regolano i poteri del Capo dello Stato e ha spiegato bene per quali ragioni in quel Paese non è vero che i poteri del capo dello Stato sono limitati, ma che invece, come in Italia oggi, il Capo dello Stato ha effettivamente una serie di prerogative. Torniamo sempre però alla stessa discussione dato semplicemente dai poteri del Presidente della Repubblica e dalla cosiddetta fisarmonica, che nel nostro Paese si apre e si chiude a seconda del contesto. Il punto particolarmente grave di questa riforma e anche la totale differenza con il modello tedesco è che qui si immagina una riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica a vantaggio del Presidente del Consiglio eletto dal popolo. Nel sistema tedesco la fisarmonica è chiusa esattamente perché quelle prerogative sono costituite sulla base del sistema dei partiti che rappresenta in quel Paese l'elemento di stabilità.

il principale partito di opposizione nel 2007, il MoVimento 5 Stelle nel 2009, Sinistra Italiana SEL nel 2010.

i cristiano-democratici e i liberali sono nati subito dopo la guerra nel 1945 ed esistono ancora; poi certamente anche in Germania ci sono partiti nuovi o almeno più recenti, come la Linke, che è nata nel 2007, e il partito di destra radicale Alternative für

la prerogativa di quel sistema è quella di essere tutto centrato su questo, cioè quel modello ha definito degli elementi di stabilità per cui anche i poteri del Presidente della Repubblica, quando la fisarmonica è stretta, sono però determinati esattamente sulla robustezza del sistema dei partiti. In questo caso, però, si ragiona su un modello che non c'entra nulla con quello, quindi non tiriamolo in ballo in maniera a mio avviso completamente sbagliata. Il sistema istituzionale che avete in mente voi non solo riduce i poteri del Presidente della Repubblica (questo è il punto), ma lo fa a favore di un sistema di partiti rinnovato, oppure a favore del Presidente del Consiglio eletto dal popolo in maniera maggioritaria e plebiscitaria? Questa è la domanda di fondo e secondo me è la cosa che proprio non funziona

vorrei però che si discutesse di una cosa così seria, cioè dei poteri del Presidente della Repubblica, esattamente in relazione al sistema istituzionale di cui si sta parlando mi spaventa molto che quelle prerogative e quei poteri vengano messi in discussione non a vantaggio del sistema democratico dei partiti, ma di un'unica persona: il Presidente del Consiglio eletto dal popolo, che quei poteri li accentra totalmente nelle proprie mani, a mio avviso con un elemento di stortura davvero molto pericoloso. Pertanto, per favore, se dobbiamo fare un ragionamento, cerchiamo di farlo in maniera seria, altrimenti facciamo anche una figuraccia con gli altri Paesi europei che penseranno che nemmeno nel diritto comparato riusciamo a dire cose che hanno qualche elemento di fondamento.

c'è un tema gigantesco che ci trascineremo per decenni come elemento di sistema. La destra vuole introdurre in Costituzione un premio di maggioranza elettorale e vuole farlo nel momento stesso in cui trasforma, di fatto, il nostro sistema da parlamentare come è adesso, come lo hanno voluto i nostri Padri costituenti a garanzia della libertà e della partecipazione, in un sistema di di fatto presidenziale, in un presidenzialismo accentuato, esasperato, dove il Presidente è il Capo del Governo eletto direttamente. Nessuno, nemmeno lei, signora Ministro - la prego di ascoltare - può negare

della nostra democrazia. Tutto questo è, nei fatti, una minaccia per la nostra democrazia liberale, che voi dite di voler sostenere e che invece qui, con presunzione e con protervia, volete conculcare, con questa legge che minaccia i fondamenti della nostra democrazia: da una parte perché è un "presidenzialismo" senza contrappesi e dall'altra perché è di fatto una legge elettorale che sarà truffaldina nei confronti dei cittadini, perché non potrete impedire che ci siano più di due candidati alla carica di Capo del Governo e quindi con un riscontro elettorale molto inferiore a quella soglia del 40 per cento invocata dalla Corte costituzionale, che voi sempre citate. Vi sarà un premio di maggioranza abnorme e truffaldino. Fate questo perché guardate esclusivamente al vostro interesse immediato. Invece la Costituzione è di tutti dovreste ragionare di princìpi, non per convenienza del momento. Fate una riforma per gli appetiti dei capi di turno, di Meloni, di Salvini, ma questo non ha niente a che fare con gli interessi dei cittadini. Serve invece una riforma una riforma nell'interesse dei cittadini. C'è un grande inganno nel vostro *slogan* «decidi tu»: una volta che il cittadino avrà scelto il Capo del Governo, poi non conterà più nulla, perché voi state portando all'estremo i mali del sistema attuale. Negli ultimi trent'anni la personalizzazione, la gerarchizzazione del sistema non sono stati un bene, signora Ministro, al contrario! I cittadini oggi hanno meno potere rispetto a trent'anni fa, perché c'è solo un modo per rafforzare le prerogative dei cittadini ed è la partecipazione, il ruolo delle associazioni, i ruoli di partiti come libere associazioni e come soggetti che costruiscono la democrazia. Signor Presidente, concludo ricordando i due articoli cardine della nostra Costituzione: l'articolo 2, che prevede la Repubblica «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; l'articolo 3, che conoscete, per il qualeè compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, l'eguaglianza, partecipazione, il pieno sviluppo della persona umana, impediscono la realizzazione e il progetto di vita di ognuno. Con questa vostra "riforma", con questa vostra concentrazione esasperata, con questa gerarchizzazione esacerbata, voi impedite tutto questo. Voi ingannate i cittadini per un vostro calcolo di potere. di potere. Ma questa iattura, questa protervia, sarà uno sfregio per la nostra società, per la nostra Repubblica, per la nostra Costituzione e si ritorcerà contro tutti. Per questo, facciamo appello ad una grande mobilitazione per impedire tutto questo. dichiarazione di voto.

È la possibilità che il *Premier*, quando doveva venire in Senato a sottoporre il proprio pensiero e la propria azione, avesse paura temesse le Camere. Temeva la Camera dei deputati, poi doveva venire anche qui. Temeva i senatori, temeva i deputati. Doveva venire alle Camere e sottoporsi al giudizio al giudizio dei rappresentanti del popolo. Poteva avere anche un'idea e, al limite, poteva anche cambiarla, respirando ciò che respirava nelle Aule: è vero o no? Quante volte abbiamo visto qui Presidenti del Consiglio presentarsi terrei in volto. Si giocavano parte della loro sorte al Governo, passando attraverso le Camere. Signora Ministra, lei ricorderà quante sedute convulse ci sono state e la tensione che si respirava. Con questo articolo, Ministro, finisce tutto. Con questo articolo, lì comparirà la parola applausi. Sarà un trionfo del Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio verrà qui a parlare alla sua tifoseria, alle persone che gli devono tutta la gratitudine e al quale sono legati. Sarà una cavalcata meravigliosa! Anzi, quando avrà difficoltà politica, correrà immediatamente in quest'Aula, perché qui saremo pronti ad applaudirlo,

perché ha preso la parola e perché ha provato a replicare a considerazioni che noi abbiamo fatto. Signora Ministra, mi lasci però dire che le sue repliche non hanno apportato al confronto alcun contributo; non se ne abbia. Quando vogliamo Quando vogliamo far vivere il confronto per davvero, abbiamo due tipi di argomenti. Abbiamo gli argomenti di valore, e su questo terreno, al momento, le distinzioni tra la maggioranza e il Partito Democratico sono abissali e inconciliabili. Si può ritenere, come come voi ritenete, che sia preferibile vivere in un ordinamento nel quale il potere è concentrato: questo è il senso della riforma. Voi proponete un modello di istituzioni nel quale il potere si concentra in una sola persona. Noi riteniamo che sia preferibile invece vivere in un ordinamento nel quale il potere è diviso, separato e limitato. Non le voglio ricordare il famoso articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, però forse varrebbe la pena tenerlo a mente, signora Ministra. Questo famoso articolo 16, che a volte anche lei mi sembra volesse volesse ricordare, recita: «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione». La Costituzione è infatti è separazione e limitazione del potere. Su questo terreno noi ci saremmo aspettati argomenti che spiegassero come i cittadini, a vostro giudizio, potrebbero vivere meglio; come i cittadini potrebbero sentire aumentate le loro possibilità di realizzazione in un ordinamento nel quale il potere è concentrato. Noi in Commissione e in Aula abbiamo cercato di spiegare perché un ordinamento nel quale è garantita la separazione dei poteri sia un ordinamento nel quale i cittadini sono più liberi e ci sono più condizioni di crescita e di sviluppo per l'intero Paese. La libertà, la separazione del potere, la garanzia dei diritti, a nostro giudizio, non sono solo una fondamentale condizione per rispettare la primazia della persona, ma sono anche una condizione di crescita e di sviluppo. qui siamo sul terreno dei modelli di convivenza che sono preferibili. E a questo riguardo voi non avete speso una sola parola per spiegare, ripeto, le ragioni per cui sarebbe preferibile uscire dalla tradizione del costituzionalismo e imboccare la strada della concentrazione del potere, quindi della primazia del Governo sul Parlamento.

oltre e dopo aver argomentato sul piano dei valori e registrato, ripeto, una distanza al momento incolmabile tra voi, la destra e questo Governo, e l'idea che abbiamo noi di democrazia e di pluralismo, abbiamo anche cercato di mettere in luce alcune contraddizioni, alcune aporie. Quella relativa alla legge elettorale e al come garantire contemporaneamente premio di maggioranza e principio di rappresentatività, lei, signora Ministra, non ha risposto. Non ha risposto lei, non ha risposto prima di lei il relatore, non ha risposto il senatore Lisei, perché la risposta da un punto di vista logico è impossibile. Prendete atto del fatto che su questo terreno, come sul terreno del merito, non avete argomenti

alla luce dell'attuale testo costituzionale, così come approvato dalla Commissione, il Parlamento, i senatori e i deputati, saranno eletti non solo in conseguenza del

l'elezione a strascico non c'è perché non c'è ancora la legge elettorale? Io penso che lei non volesse intendere questo quando ha risposto con queste parole. Io penso che lei avesse ben altre considerazioni. Allora queste altre considerazioni, per cortesia, ce le dica e ci faccia partecipi di come il Governo intende risolvere questo secondo ordine di considerazioni di carattere logico e giuridico, non considerazioni di merito sul quale purtroppo, insisto, non avete...

quella legata alla costituzionalizzazione della legge elettorale che andrebbe invece trattata con legge ordinaria e l'assenza della soglia. La modifica introdotta con l'articolo 6 di questo provvedimento all'articolo 57 della Costituzione rappresenta un effetto collaterale della costituzionalizzazione della legge elettorale. È un errore da correggere, nel senso che prevedere che il premio di maggioranza alla coalizione collegata al Presidente eletto sia corrisposto su base nazionale, all'interno di una legge che invece, per diversa previsione costituzionale, non comporta l'assegnazione nazionale di seggi, ma l'assegnazione regionale, l'assegnazione regionale, significa violare il principio di coerenza e omogeneità interno alla legge elettorale stessa, nazionale di seggi laddove invece l'assegnazione oggi è regionale e stiamo portando avanti un premio di maggioranza alla coalizione collegata al Presidente eletto su base nazionale. Cioè da un lato c'è la base nazionale, dall'altro c'è l'assegnazione dei seggi su base però il meccanismo rimane nazionale. Quindi, come minimo, alla previsione di un premio di maggioranza nazionale avrebbe dovuto corrispondere una modifica dell'articolo 57 con il superamento del criterio regionale di assegnazione dei seggi. Qui non stiamo parlando di ideologia o di posizioni politiche differenti; stiamo parlando di un errore che deve essere corretto. Diversamente incorriamo in un principio di incoerenza della legge elettorale. Almeno questa questione, che è tecnica e non politica, la volete prendere in considerazione e provare a metterci una pezza, sì o no? Questa è la nostra richiesta.

sia sterile e che noi dell'opposizione ci stiamo limitando a ripetere più o meno sempre quei due o tre concetti, semplicemente per riempire uno spazio temporale. Invece io vi garantisco, cari colleghi e care colleghe, Presidente, Ministra, che non è affatto così, perché più si ha l'opportunità di riflettere, di analizzare e anche di ascoltare i contributi degli altri e delle altre e più davvero questo testo, che voi sottoponete *coram populo*, perché, sottoponendolo in quest'Aula, lo affidate anche alla lettura e all'intelligenza degli italiani e delle italiane, è inspiegabile. È un testo la cui origine è assolutamente inspiegabile. Avete cominciato con un testo snello, che agiva su quattro articoli della Costituzione. E ve ne siete vantati, dicendo: modifichiamo soltanto quattro articoli della Costituzione, è una modifica minimale, una modifica non invasiva, perché l'importante per noi è raggiungere l'obiettivo della governabilità. Poi vi siete resi conto che era un assurdo quello che stavate dicendo e quindi avete dovuto cominciare ad aggiustare anche quell'altro articolo e quell'altro ancora; avete dovuto prendere quell'altro articolo ancora. Vi siete resi conto che quello che volete raggiungere è impossibile è impossibile senza stravolgere la Costituzione nel profondo. Perché dico questo? Perché noi stiamo votando l'articolo 6, che è minimale. Cosa fa Aggiunge all'articolo 57 della Costituzione, dove si stabilisce come si vota il Senato della Repubblica, «e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92». Ossia vi state incaprettando mani e piedi. Prima Prima qualcuno ha detto che avete avuto la faccia tosta di dire che non avete voluto collegare una legge elettorale all'interno della Costituzione, negando anche qui una realtà palese. Voi avete inserito il premio di maggioranza in Costituzione; questo è il motivo per cui poi vi siete accorti che dovevate modificare anche l'articolo 57, perché state apportando uno sfascio totale, da cui non sapete più neanche voi come uscire. Io mi sto convincendo, attraverso questa lunga discussione, che non è stata inutile, che voi questa riforma ve la rimangerete e non avrete il coraggio di sottoporla alla Corte costituzionale per un *referendum* costituzionale, perché è un obbrobrio senza capo né coda. È una cosa giuridicamente impresentabile ed è davvero la spia che denuncia la vostra pura sete di potere. Razionalmente non si spiega un pastrocchio del genere, che vi sta costringendo a correggere voi stessi, a tornare su quanto avete scritto, ad aggiustare. Non ci avete detto come i 5 milioni di italiani all'estero come i 5 milioni di italiani all'estero eserciteranno il loro diritto costituzionale di essere uguali agli altri elettori, sfasando potenzialmente e completamente il peso del voto sull'elezione del *Premier*. Non ci avete detto come gli italiani si recheranno alle urne, quante croci dovranno mettere, quante schede avranno. Vi siete infilati in un vicolo cieco. È per questo che sono sicura - a questo punto sto maturando la convinzione - che questa roba

Condivido con la Ministra l'idea che questa discussione sarebbe dovuta avvenire in modo diverso, più costruttivo e più condiviso. Fatico tuttavia a comprendere perché si scarichi sull'opposizione la responsabilità di questa modalità che ci ha costretti all'ostruzionismo. Certamente, infatti, non è un dialogo costruttivo, quello della convocazione una volta soltanto

A casa mia l'interlocuzione e il dialogo avvengono in maniera diversa; non solo convocando per ascoltare l'opinione degli altri, ma anche provando a misurarsi sull'esistenza di un terreno comune di intesa e di possibile riforma.

per cui la riforma se la fanno in casa e, o la va o la spacca, si va al *referendum* senza tentare un approccio dialogante con le opposizioni. Inviterei la maggioranza a tener conto delle parole che ha pronunciato oggi il cardinal Zuppi, che ha detto che la nostra Costituzione fu il frutto di un'alta condivisione di ciò che univa e fu scritta grazie al contributo delle maggiori culture del Paese, socialista, comunista e liberale. È buon senso - ha detto il cardinal Zuppi - usare per le riforme quello riforme quello stesso inchiostro, cioè l'inchiostro di una condivisione. Cosa che invece purtroppo non avviene. Io sono però fiducioso

sarebbero ancora praticabili. L'articolo 7 su cui stiamo ragionando e su cui ho presentato un emendamento è, secondo me, la *summa* di tutte le contraddizioni di questa riforma. In tale articolo si prevede infatti che il *Premier* eletto direttamente dai cittadini debba avere anche la fiducia delle Camere.

un *Premier* è eletto direttamente dai cittadini, che bisogno ha della fiducia del Parlamento? E allora cosa fate voi per garantire che non ci siano contraddizioni tra un *Premier* eletto dai cittadini che non ha la maggioranza e quindi la fiducia del Parlamento? coartate la rappresentanza parlamentare, attraverso quel sistema di elezione contestuale al *Premier* eletto direttamente dai cittadini (elezione a strascico, a rimorchio, chiamatela come volete), e scrivete addirittura in Costituzione che la legge elettorale deve deve garantire la maggioranza al *Premier* eletto, in questo modo stravolgendo i principi posti dalla Corte costituzionale che riguardano la rappresentanza. Infatti, in un

coartata in funzione della maggioranza che deve essere data al *Premier,* state semplicemente abbandonando il sistema parlamentare che dite di voler garantire e salvaguardare. Questa è una contraddizione che voi non siete in grado di risolvere, perché nessuna legge elettorale può garantire la maggioranza al *Premier* eletto direttamente dai cittadini, salvo una legge elettorale che rende non più rappresentativo il Parlamento, perché a quel punto anche una maggioranza del 30 per cento dovrà essere trasformata in una maggioranza di oltre il 50 per cento. Questo è il nodo, perché a quel punto il Parlamento non sarà più rappresentativo, il sistema parlamentare non ci sarà più, perché diventa di fatto un sistema presidenziale, con tutte le conseguenze che si porta dietro, perché un Parlamento eletto in questo modo sarà anche quello che elegge il Presidente della Repubblica con quella stessa maggioranza; inoltre il Presidente della Repubblica elegge cinque giudici della Corte costituzionale

Queste sono le ragioni per le quali noi ci opponiamo così strenuamente, non per un pregiudizio, ma perché vediamo tutti i rischi di questa architettura istituzionale che state immaginando e vi invitiamo ad abbandonarla per trovare i terreni d'intesa possibili, che ci sono se solo voleste provare a ragionarci insieme.

vorrei, sempre tramite lei, rivolgermi alla Ministra, che naturalmente in queste occasioni ha molto da telefonare, ma è importante che tra una telefonata e un'altra ci ascolti, soprattutto quando noi ci riferiamo a quello che lei ha detto. ha detto e ha ripetuto che non capisce e si meraviglia del perché, rispetto alle poche risposte che abbiamo alle nostre domande, noi reagiamo ribadendo le stesse domande. Io le vorrei dire che questo capita, in genere (non solo in politica, non solo in questo dibattito), quando le risposte non rispondono alle domande. se lei mi rivolge una qualunque domanda e io rispondo parlando d'altro, immaginando di aver ascoltato una cosa che non è quella che mi ha chiesto, lei reagirebbe come chiunque di noi, ribadendo quella domanda. Le assicuro che è esattamente la regola che sta alla tesi, antitesi e sintesi: la sintesi può esserci se le due tesi sono sullo stesso piano. Le assicuro che sarebbe d'accordo anche Hegel. Dopo che il presidente Gasparri ha chiamato il re Carlo, voi potete mandare anche un messaggino WhatsApp a Hegel, ve lo confermerebbe. Se le due tesi sono su piani diversi, non ci può essere alcuna sintesi. alcuna sintesi. Il fatto che non ci sia un dialogo e che anche le risposte che abbiamo ascoltato siano state risposte non alle nostre osservazioni e domande è dimostrato da tutti gli esempi che sono stati fatti di diritto costituzionale comparato. Io, per mio limite, non ho mai capito se i riferimenti che sono stati fatti a Francia, Germania e Inghilterra erano per dire che questa vostra riforma ha degli esempi altrove, oppure che si fa il contrario rispetto ad altri sistemi istituzionali. Abbiamo ascoltato i riferimenti all'Inghilterra per dimostrare che non è vero quello che si dice a proposito del premierato, per poi dire, però, che in Inghilterra non si elegge direttamente il Primo Ministro. La Ministra qui ha detto che il Parlamento francese non conta, ora ha anche aggiunto che il Presidente della Repubblica tedesca non conta niente. Naturalmente faccio sempre notare che siamo nell'Aula del Senato della Repubblica italiana e non al dopolavoro ferroviario; non so se questa sia la posizione del Governo, perché io ho ripetuto parole testuali: "il Parlamento francese non conta, il Presidente della Repubblica tedesca non conta". Altre volte si è invece citata la Francia per dimostrare che anche lì il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e non è che lì non vi sia la democrazia. Non ho mai capito se questi esempi servissero per corroborare la tesi di questa riforma o per metterla in contraddizione. Di certo c'è che viene proposto non c'è da alcuna parte al mondo. *(Applausi).* Si rivendica il fatto che questa è una riforma all'italiana. Va bene, sarà che gli altri non hanno avuto il genio italico che adesso si concretizza in questa riforma,

è già stato fatto altrove. Mi tocca far notare che quando c'è un dialogo con il Governo i parlamentari, anche quelli più autorevoli, devono rispettare gli altri parlamentari che parlano. ascolti, non è corretto che lei dica che noi non abbiamo fatto proposte, perché dal primo giorno, prima ancora che fosse scritta una sola riga, quando lei ha incontrato la delegazione del Partito Democratico, ha ricevuto una nostra proposta puntuale, che peraltro esiste in natura, cioè l'abbiamo avanzata e abbiamo dimostrato che altrove funziona. D'altra parte, lei parlava prima con il senatore Pera, il in questo dibattito, non da questa parte dell'Aula, ha indicato aporie e contraddizioni; se anche voi avete indicato in questo stesso testo che state votando acriticamente aporie e contraddizioni, emendatelo e modificatelo, altrimenti state portando avanti non un dialogo, non un confronto, nemmeno con voi stessi; non riconoscete nemmeno i vostri stessi limiti. Ministra, lei ha ripetuto ancora una volta che siete partiti dal presidenzialismo e siete arrivati a questa proposta per venirci incontro. Ebbene, noi le ripetiamo ancora una volta che questa proposta è più lontana dalle nostre di quella che avete Presidente. Non so come dirlo meglio, non perché il premierato sia più lontano, ma perché questo ircocervo è più lontano. Sarebbe stata, per quanto non l'avremmo condivisa, più logica la proposta che avete fatto agli italiani con il presidenzialismo.

diverse leggi elettorali possono essere coerenti, ma ci deve pur essere una gamma, altrimenti anche questa proposta diventa monca. Concludo dicendo che non convincerete mai gli italiani. Il presidente Romeo ha detto chiaramente che c'è un patto: il presidenzialismo, l'autonomia differenziata e la riforma della giustizia. Non convincerete mai gli italiani che l'esigenza che loro hanno sia di far fare a Giorgia Meloni e a questo Governo quello che il Parlamento gli impedisce, perché non gli stiamo impedendo niente; quello che i senatori a vita gli impediscono, perché non gli stanno impedendo niente; quello che il Presidente della Repubblica gli impedisce, perché non gli sta impedendo niente.

dell'opposizione. In particolare, vorrei replicare al collega Bazoli che non è affatto vero che la fiducia al Governo prevista da questo articolo articolo sia in contraddizione con l'elezione diretta del *Premier*, perché certamente a lei non è sfuggito che un conto è il Presidente del Consiglio, un conto è il Governo. Noi prevediamo, certo, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma questo non toglie che, nel momento in cui il Presidente del Consiglio forma il Governo, sia giusto un passaggio parlamentare, affinché il Governo nel suo complesso abbia la fiducia del Parlamento, proprio per valorizzare il ruolo del Parlamento nella formazione del Governo e per non fuoriuscire da quel modello parlamentare o neoparlamentare cui lei faceva riferimento. Non è vero, come ho cercato di spiegare in altra occasione, che il Parlamento non sia più rappresentativo perché è previsto un premio di maggioranza per il *Premier* eletto:

della composizione complessiva del Parlamento. Se fosse vero il suo ragionamento, collega, allora dovremmo concludere che anche tutte le Assemblee legislative delle Regioni non sono rappresentative. Sono assemblee legislative anche quelle, eppure anche lì vige il principio per cui il Governatore che vince trascina un premio di maggioranza; per non parlare dei Comuni, dove addirittura il premio è pari al 60 per cento; e per non parlare dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, dove addirittura il premio è pari al 66 per cento. Qui noi, ovviamente, immaginiamo un premio enormemente più ridotto di questo. Tra l'altro, ho fatto già in quest'Aula negli scorsi dibattiti un esempio, citando i risultati

Sapete, colleghi, qual è l'unico caso nel quale si sarebbe dovuto ricorrere al premio di maggioranza? L'unico caso, su 10-12 Regioni in cui si è votato, nel quale si sarebbe dovuto ricorrere al premio di maggioranza è, guarda caso, la Sardegna: l'unico caso in cui, applicando il principio del premio di maggioranza, c'è stato bisogno di ricorrere a questo premio è stata la Sardegna. Non vi dice niente che in Sardegna il centrosinistra avrebbe perso, se non si fosse applicato il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione, perché sulla base delle liste, il centrosinistra è arrivato sette punti percentuali dietro? Questo a dimostrazione del fatto che la democrazia diretta può essere anche un valore, persino per il centrosinistra. Al collega Fina, che lamenta che non c'è stato il dialogo, dico: certo, fra due parti che rifiutano di ascoltare l'altra il dialogo è difficile che ci sia; soprattutto, è impossibile che si arrivi alla sintesi. Non è che la maggioranza non ascolti l'opposizione; semplicemente, la maggioranza e il Governo ascoltano l'opposizione, ma purtroppo un limite nostro o un limite vostro. Non so, giudicheranno gli italiani, perché alla fine saranno loro a pronunciarsi con un *referendum* su questa riforma. Spero almeno che siamo tutti d'accordo che sia giusto, legittimo, doveroso e sacrosanto che alla fine siano gli italiani a dire se questa riforma va bene o non va bene, se vogliono scegliere direttamente il *Premier* con il loro voto o se vogliono affidarsi ancora alla mediazione dei partiti. Questo è giusto che siano gli italiani a dirlo. Collega Fina, non è che siamo noi che non ascoltiamo voi; siete voi che non riuscite a convincerci. Faccio solo un esempio, visto che continuate a invocare il sistema tedesco. Ebbene,

sulla sfiducia costruttiva, siamo d'accordo su questo? La sfiducia costruttiva prevede che il Bundestag, se decide di cambiare un Cancelliere, gli deve votare la sfiducia e deve indicare nella mozione mozione chi gli deve subentrare. Mi sapete dire qual è il margine di discrezionalità e qual è il ruolo che svolge in questo contesto il Presidente della Repubblica federale tedesca? In altri termini, potrebbe il Presidente della Repubblica federale tedesca nominare Cancelliere una una personalità diversa da quella il cui nome e cognome sta scritto nella mozione di sfiducia costruttiva? Certamente non potrebbe, perché farebbe un attentato alla Costituzione. Siamo d'accordo su questo? Allora la domanda che vi faccio è molto semplice, colleghi dell'opposizione: perché non va bene se il vincolo deriva direttamente dal popolo che detiene la sovranità popolare, mentre se mentre se deriva dal Parlamento allora va bene? Penso che debba andare bene in entrambi i casi. Il sistema tedesco ha le sue regole, mentre noi ci scriviamo le nostre. Non ci sono esempi - dite voi che collimano con le regole che noi stiamo proponendo. È vero. Vi faccio semplicemente e rispettosamente notare che neanche in Francia c'erano precedenti prima che De Gaulle si inventasse la Repubblica semipresidenziale, e la la sinistra di allora gridava, esattamente come fate voi adesso, al pericolo fascista e autoritario, nonché allo stravolgimento della democrazia, e delle regole dello Stato di diritto esattamente come fate voi adesso). Sapete fino a quando? Fino a quando Mitterrand ha vinto le elezioni presidenziali francesi: da quel momento in poi, la Repubblica presidenziale francese anche per la sinistra francese è diventata un modello straordinario da sottoscrivere. Colleghi, da questo punto di vista, mi sembra di aver spiegato ampiamente perché come relatore esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 7, tranne all'emendamento all'emendamento 7.900 del Governo, perché certamente riscrive in modo più chiaro e ancora più inequivocabile le regole con cui si dovrà procedere in caso di dimissioni, di morte o di impedimento del Presidente del Consiglio. Ringrazio da questo punto di vista il Ministro per il lavoro di

scoprirete che vi si cerca di dare risposta anche ad alcune delle osservazioni che avete avanzato in Commissione e anche in Aula, proprio a dimostrazione del fatto che non è vero che non ascoltiamo e, quando ci sollevate questioni ragionevoli, anzi le accogliamo,

vorrei soffermarmi su questa riformulazione dell'articolo 7, perché la riforma introduce per la prima volta una regolamentazione di tutte le crisi di Governo, definendo e disciplinando anche le possibili soluzioni. Sono le forze politiche che devono assumersi la responsabilità di fronteggiare le varie tensioni e lo devono fare proprio per preservare la figura del Capo dello Stato e la sua autorevolezza,

lo sappiamo tutti e lo diceva acutamente anche il costituzionalista Cassese, era costretto a dilatare la fisarmonica dei suoi poteri ogniqualvolta il sistema parlamentare non funzionava. Quindi non possiamo rassegnarci a trovarci sempre di fronte a crisi che destabilizzano il nostro sistema e considerarle come un carattere permanente del nostro sistema

dei poteri e di pesi e contrappesi dei vari ruoli istituzionali. Quando parlo di pesi e contrappesi, penso al rapporto tra Governo e Parlamento, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. siccome si dice che con questa regolamentazione andiamo a limitare le occasioni in cui il Capo dello Stato interviene nelle varie crisi, l'osservazione è appunto quella che il Capo dello Stato mantiene tutte le sue prerogative e, stabilendo le possibili soluzioni delle crisi,

dell'unità, come rappresentante dell'unità nazionale, dall'altro, il Presidente del Consiglio ha un ruolo di indirizzo politico. Tali ruoli non possono e non devono mai sovrapporsi.

vorrei chiarire, anche al presidente Balboni, che non è l'opposizione che non vuole il dialogo. Anzi, lo sta sollecitando: più volte, in Commissione e in quest'Aula, ho continuato a chiedere al Ministro di darci una spiegazione sola: la compatibilità di questa riforma con lo Stato di diritto e con il bilanciamento dei poteri. Non c'è stata risposta e forse a questo silenzio un significato dovremmo pure darlo. Questa volta voglio leggere, perché mi sembra che siano risultate inutili le mie parole. Mi rivolgo di nuovo ai colleghi giuristi. Partiamo da cose più semplici: la definizione dello Stato di diritto.

nel diritto è uno dei principi giuridici fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia liberale. al sito della Commissione europea. Vi leggo queste due righe e vi pregherei di ascoltare; lo chiedo in particolar modo ai colleghi giuristi. Si legge che lo Stato di diritto è uno dei valori fondamentali dell'Unione, lo sancisce l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, ed è anche la *conditio sine qua non* della tutela di tutti gli altri valori fondamentali dell'Unione, a cominciare dai diritti fondamentali e dalla democrazia. Il rispetto dello Stato di diritto è capitale per lo stesso funzionamento dell'Unione - ascoltate - efficace applicazione del diritto dell'Unione, corretto funzionamento del mercato interno, mantenimento di un contesto propizio agli investimenti. Colleghi, sapete di cosa stiamo parlando? C'è un'infografica, sempre nel sito del Parlamento europeo, che parla di questi valori e che ribadisce come valore condiviso lo Stato di diritto. Parla di valori fondamentali e li mette alla stessa stregua della dignità umana, che voi spesso dimenticate quando si parla di salario minimo, quando si fa un trattamento disumano dei migranti. Parlano tutti di questo. Mi sono voluto togliere una curiosità. Vediamo cosa succede andando su un sito del Governo. Mi sono collegato con il sito C'è su Google un risultato sullo Stato di diritto dell'Unione europea, quello su cui voi non rispondete. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Apro la pagina, la connessione non è privata, non c'è scritto più nulla. Allora quantomeno, Ministro, ce la vuole dare lei una risposta? Com'è compatibile con lo Stato di diritto quest'obbrobrio di diritto costituzionale?

espresso parere negativo e la maggioranza ha espresso un voto sempre contrario. Servivano soltanto a denotare e a caratterizzare i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, che di fatto la vostra riforma, che stiamo affrontando in queste ore in Aula,

non può neanche nominare direttamente i Ministri o revocarli. Lo deve fare sempre per il tramite del Presidente della Repubblica e questo non per la volontà di salvaguardare il ruolo e le prerogative del Presidente, ma per l'approccio che il

che continua a voler andare avanti con questa riforma costituzionale, ma si ostina a dire che la sua riforma è fatta con piccoli e leggeri colpi di penna che vanno a tagliare qua e là qualcosa, ignorando o volendo ignorare, nonostante quello che abbiamo detto più volte, che una riforma di questo genere doveva essere accompagnata da una intera revisione del nostro assetto parlamentare non per stravolgere i poteri, ma per armonizzarli. Se c'era un'equazione che in questo momento comunque aveva funzionato, nel momento in cui andiamo a cambiare gli elementi, dovremmo anche

non è più così: non è più un organo collegiale, giacché vogliamo eleggerlo direttamente. È perciò incomprensibile la ragione per la quale è stato un parere contrario da parte del relatore e del Governo e incomprensibile è altresì tutto l'approccio che è stato adottato nei confronti degli emendamenti e delle proposte che ha formulato Italia Viva.

magari *re melius perpensa*, se ci fosse stata un'apertura in Aula, saremmo stati ben lieti di accoglierla. Così però non è stato. Non è stato su tutto quello che abbiamo chiesto di modificare e sugli interventi che andavano fatti sugli istituti repubblicani per garantire veramente che questa riforma funzioni. Voi ci avete detto sempre di no, ostinatamente di no e io direi anche immotivatamente di no. Su questo emendamento continuo a ribadire l'importanza di un confronto serio, reale e concreto

che il potere appartiene sempre al popolo e per questo ci batteremo sempre. Nel momento però in cui si creano un'occasione di confronto e un procedimento di riforma costituzionale, si deve lavorare al meglio delle capacità per realizzarla e io ritengo che questa non sia la migliore riforma possibile. Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione di questo emendamento per replicare al presidente Balboni, che ha avuto la gentilezza di ascoltarmi e di fare alcune considerazioni sulle mie riflessioni, che peraltro non mi hanno convinto. Senatore Balboni,

lei sta dicendo che, nell'ipotesi in cui il *Premier* non dovesse raggiunge quella soglia, non scatterebbe il premio di maggioranza. Quindi, per un verso, quella legge sarebbe incostituzionale, perché voi avete detto che la legge deve garantire un premio su base nazionale che garantisca la maggioranza dei seggi nelle Camere e questa non lo garantirebbe; per altro verso, sarebbe una legge che non garantisce la maggioranza, quindi che non garantisce al *Premier* eletto direttamente dal popolo di avere la fiducia del Parlamento.

che afferma che in una forma di governo parlamentare ogni sistema elettorale, seppure deve favorire la formazione di un Governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. ad un sistema di governo parlamentare. Non si può derogare a questo principio. Forzare una legge elettorale per andare dietro all'elezione diretta del *Premier* rischia di sacrificare il valore costituzionale della rappresentatività. La Corte

dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale e quindi, secondo la Corte, è ben diverso dalla forma di Governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale. Allora delle due l'una: o volete salvaguardare la forma di Governo parlamentare, e allora non potrebbe mai farlo una legge che si accompagni all'elezione diretta del *Premier*, o altrimenti state facendo un presidenzialismo di fatto,

perché condividiamo la necessità di stabilizzare i Governi e di rendere più forte e chiaro il ruolo del Presidente del Consiglio, ma quest'obiettivo non si raggiunge con l'elezione diretta, bensì attribuendo al *Premier* veri poteri, non solo di coordinamento, ma di decisione; poteri che devono essere più simili a quelli del Primo Ministro britannico e a quelli del Cancelliere tedesco. Pertanto, pensare che l'elezione diretta del *Premier* da sola determini la stabilizzazione dei Governi e un rafforzamento dei poteri del *Premier* secondo noi non corrisponde al vero. Quello che serve

Signora Presidente, desidero rivolgermi al relatore Balboni e al Ministro, pregandoli di ripensare, da questo momento fino a quando non si voterà, il loro parere negativo sull'emendamento 7.900/54 a mia firma. La motivazione che mi spinge è una questione di chiarezza linguistica. La situazione è la seguente. Il Presidente del Consiglio che decide di dimettersi Il Presidente del Consiglio che decide di dimettersi si presenta al Parlamento e annuncia le sue dimissioni. Questa si chiama parlamentarizzazione della crisi: è una grande conquista, perché non è mai successo così, salvo per un caso, che il Governo sia caduto in Parlamento. Una volta fatta l'informativa al Parlamento, il Presidente del Consiglio ha sette giorni per recarsi dal Presidente della Repubblica e fare le tre cose che gli sono consentite:

credo che la successione che ha in mente il Governo sia l'informativa, che è parlamentarizzazione, e poi decisione entro sette giorni di andare dal Presidente Repubblica e fare la richiesta. Nel testo del Governo questa «Negli altri casi di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere Scritta così com'è, alla lettera, sembra che la previa informativa parlamentare riguardi lo scioglimento del Parlamento e non è questo il caso, non è questo che vuole il Governo, non è questo che dice il testo: l'informativa parlamentare riguarda le dimissioni del Governo, le ragioni delle dimissioni. Dopodiché, avendole illustrate al Parlamento, il Presidente del Consiglio ha sette giorni per andare dal Presidente della Repubblica

e non le ragioni e le motivazioni della crisi, ho riformulato queste poche righe - è una riformulazione linguistica, ma evita l'ambiguità - come segue: «Nel caso di dimissioni volontarie, da presentare al termine di una informativa parlamentare, nel caso di dimissioni dovute a reiezione di una questione di fiducia, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni» ha la facoltà di. Così è più chiaro che l'informativa riguarda le ragioni della crisi e delle dimissioni

si estenda allo scioglimento, la qual cosa comporterebbe grande confusione perché non sta al Parlamento chiedere lo scioglimento e neanche al Governo annunciarlo al Parlamento. Poiché questa riformulazione che ho fatto a me pare molto più chiara e a me pare che non cambi la sostanza di ciò che il Governo ha in mente, prego da qui a quando voteremo questo subemendamento Governo e il relatore di ripensare il loro parere contrario, perché l'emendamento ha proprio lo scopo di rendere chiaro ciò che loro hanno esattamente in mente, cioè la successione, la scansione delle fasi: informativa sulla crisi,

desidero intervenire a sostegno di questo emendamento e di altri emendamenti che abbiamo presentato, perché se l'articolo 5 è il cuore della riforma, come abbiamo detto, penso che l'articolo 7 dimostri fino in fondo quanto questa riforma svuoti di senso il Parlamento, perché ridisegna il rapporto di fiducia in modo tale, irrigidito in una serie di automatismi che vengono riproposti ulteriormente nell'emendamento che il Governo ha presentato,

Non è possibile, infatti, parlamentarizzare le crisi, non è possibile qui dentro cercare una risposta diversa, una volta che abbiamo legato, nell'articolo 5, l'esistenza stessa del Parlamento, al di là di quale sarà la soglia soglia del Parlamento, all'elezione del *Premier.* È davvero un mondo capovolto: un Parlamento al servizio del Governo, un Parlamento al servizio della maggioranza. Quello che il Presidente del Consiglio può decidere, come dimostrano anche gli interventi del relatore e del Ministro spiegando il giudizio negativo su tutti gli emendamenti presentati, è di sciogliere il Parlamento. Questo è un grandissimo potere e tale potere è tolto al Presidente della Repubblica. Per cui non è vero, come vi siete ostinati a dire, che questa riforma non ridisegna le competenze e i poteri del Presidente. E non è vero che questa riforma non svuota il senso del lavoro che noi stiamo facendo qui. Mi faccia anche dire, signor Presidente, che è sbagliato confrontare quello che noi facciamo qui, il ruolo che ha il Parlamento, con quello degli enti locali e delle Regioni. Noi stiamo parlando del luogo della rappresentanza del popolo italiano, dove risiede il potere legislativo, che non ha nulla a che vedere col premio di maggioranza di un Comune e con come si amministra un Comune ed un territorio. Francamente, è anche svilente e dimostra qual è la cultura istituzionale e costituzionale che sta dietro quest'idea di Parlamento e di Governo. Sostanzialmente, gli elettori e il popolo saranno chiamati, ogni cinque anni, a scegliere un *Premier* e da questo dipenderà tutta la vita istituzionale del Paese e tutta l'attività legislativa del Parlamento, che sarà che sarà al servizio del Governo. Il fatto che la crisi di quel Governo e le possibili dimissioni del Presidente del Consiglio determinino la vita o meno del Parlamento, con tutta la procedura che è descritta e irrigidita, io non credo darà maggior stabilità perché porterà dentro le istituzioni la conflittualità e l'instabilità e impedirà di cercare soluzioni e condivisioni. Non vi è solo la tesi e l'antitesi,

voi il Parlamento non è il luogo della relazione e del dibattito e della ricerca di soluzioni più avanzate. Questa è la morte della democrazia parlamentare. Non so definirlo diversamente.

altri a mia prima firma, perché la formulazione dell'articolo 7 - è per questo motivo che abbiamo presentato tali emendamenti - pone diverse contraddizioni e rischia anche di creare problematiche di interpretazione della Costituzione. della Costituzione. Entro nel merito, signor Presidente. La questione della fiducia richiesta all'atto di presentazione del Presidente eletto e del Consiglio dei ministri nominato è già in sé una contraddizione. Che cosa succederebbe, infatti, se il capo dell'Esecutivo designato direttamente nella consultazione elettorale si trovasse nella condizione di non ottenere la fiducia delle Camere? Ci sarebbe un'opposizione e un blocco istituzionale...

se il capo dell'Esecutivo, designato direttamente della consultazione elettorale, si trovasse nelle condizioni di non ottenere la fiducia delle Camere? Ci sarebbe un'opposizione, un blocco istituzionale tra volontà popolare e potere decisionale dei parlamentari, peraltro anch'essi appena eletti? Che senso ha dunque prevedere e predisporre la richiesta di una fiducia che contiene in sé una sorta di ricatto su più livelli? Il Parlamento, per l'ennesima volta in questo disegno di legge, viene ridotto a segretario dell'Esecutivo, pena il ritornare immediatamente ad elezioni, con tutto ciò che questo comporterebbe. Inoltre, con questo emendamento abbiamo tentato di ovviare a questa situazione paradossale e anche assurda creata dalla poca perizia del Governo nello stendere la proposta costituzionale, aggiungendo l'illustrazione del programma dell'Esecutivo per dare un senso all'obbligo per il *Premier* neoeletto e i Ministri di presentarsi davanti al Parlamento, che - lo ricordiamo - nella nostra democrazia è l'istituzione che si fa veicolo della sovranità popolare, proprio perché rappresenta la pluralità, le componenti maggioritarie e le minoranze. È al Parlamento che va dato sostegno, è il Parlamento che va tutelato, non è non un individuo solo eletto, ma la coralità dei rappresentanti. Si chiama democrazia rappresentativa. Questo mi porta alla seconda contraddizione, Presidente, di natura simile a quella appena illustrata, ma riguardante ancora una volta in questa proposta di riforma costituzionale, il Presidente della Repubblica. Non si capisce che cosa questa maggioranza trova di minaccioso nella sua figura, ma sta di fatto che in quasi ogni articolo di questo disegno di legge troviamo un attacco alle prerogative del Capo dello Stato e un tentativo di svilimento delle sue funzioni.

Di nuovo, questa maggioranza relega il Presidente della Repubblica al ruolo di funzionario di segreteria, che mette in moto procedimenti apparentemente automatici su cui non ha alcuna prerogativa di controllo. È chiaro quindi che la ragione per cui negli emendamenti abbiamo proposto di aggiungere almeno la procedura di consultazione da parte del Capo dello Stato dei Presidenti delle due Camere per verificare che realmente non ci siano le condizioni per risolvere la crisi di legislatura in essere. E che dire Presidente del fantomatico secondo Presidente del Consiglio, paradossalmente non eletto in via diretta da cittadine e cittadini, nonostante il dichiarato intento principale dell'intera proposta... Rischierebbe persino di avere più poteri del primo, quello teoricamente eletto, in quanto esente da rischi di rimpasti e macchinazioni interne della maggioranza. con questi emendamenti abbiamo provato a ovviare all'inadeguatezza e mi rivolgo ancora al Governo e alla maggioranza, con speranza spero non vana: aprite gli occhi sulla pericolosa china che sta prendendo la nostra democrazia.

Signora Presidente, abbiamo appreso poco fa una notizia e, tramite lei, chiediamo un'informativa urgente, come è stata già chiesta alla Camera anche qui in Senato, del ministro della giustizia Nordio in relazione alla deposizione che stamattina al tribunale di Roma ha rilasciato il capo del DAP Giovanni Russo, sul processo che vede imputato il sottosegretario Delmastro Delle Vedove.

Al di là dei rilievi penali - starà al tribunale stabilire le responsabilità eventuali del Sottosegretario, del quale da tempo abbiamo chiesto le dimissioni - quella limitata divulgazione, il Sottosegretario, come è noto, la interpretò come un manganello da fornire al collega di partito Donzelli, che a sua volta manganellò in Aula l'opposizione con quei contenuti.

che il capo del DAP smentisca un Sottosegretario che ha le deleghe alla Polizia penitenziaria, che ha compiuto probabilmente un grave reato. Se ne deve andare. Nordio deve riferire.

anch'io mi unisco alla richiesta del collega Verini. Mi sembra un fatto importante, non soltanto per l'uso che poi è stato fatto di questa documentazione, ma soprattutto perché, in un momento nel quale ci occupiamo di *cybersecurity* e quindi della tutela dei dati della pubblica amministrazione, il fatto che dentro il Governo ci sia una violazione dei protocolli di riservatezza della documentazione, in particolare del Ministero di del Ministero di giustizia, ci preoccupa moltissimo. Per cui, al di là del fatto in sé, vorremmo che il ministro Nordio venisse a rassicurarci sulla solidità dei protocolli e delle procedure che sono tese a garantire la confidenzialità degli atti del Governo, perché si tratta di atti che spesso rivestono un carattere di profonda riservatezza. Se è così semplice che documenti riservati possano circolare al di fuori di quelle cerchia nelle quali devono restare per legge, questo ci preoccupa in linea più generale. politico, credo che ci sia una questione di *compliance*, che però ha a che fare con la sicurezza del Paese. Per cui terremmo molto a sentire il ministro Nordio ed eventualmente il sottosegretario alla Presidenza Mantovano, proprio per gli aspetti che hanno a che fare con la sicurezza dello Stato.

sulla richiesta del collega Verini, alla quale si sono già associati altri Gruppi dell'opposizione. Le devo dire, Presidente, che sono veramente meravigliato che un collega, che si è costituito parte civile nel processo che si è costituito parte civile nel processo nei confronti dell'onorevole Delmastro utilizzi e strumentalizzi la sua carica parlamentare e il suo ruolo in quest'Aula, che è chiaramente in totale e plateale conflitto di interessi con la sua costituzione di parte civile per strumentalizzare un'affermazione fatta da un teste nell'ambito di un processo nel quale il collega Verini vuole fare contemporaneamente la parte civile e il giudice.

Se il Presidente mi ha dato la parola, vorrei parlare.

che in democrazia si dovrebbe parlare anche quando si dicono cose che non piacciono all'opposizione. Io stavo semplicemente spiegando che, secondo il nostro sistema penale, rivelare una notizia a chi ha il diritto di conoscerla non è reato. Questo lo dice tutta la giurisprudenza, se vogliamo fare il processo qui.

che vi stavate facendo strumentalizzare dai terroristi e dai mafiosi. Questa è la verità. *(Applausi.

il presidente Balboni si è sostituito al Governo e non mi pare faccia ancora il Ministro della giustizia. *(Applausi)*. Noi abbiamo chiesto attraverso, il senatore Verini, che il Governo facesse esattamente quello

perché è costituito parte civile, è un'offesa. *(Commenti)*. È un'offesa alla verità!

*(PD-IDP)*. Signora Presidente, questa è l'ennesima dimostrazione che questa destra che sta stravolgendo la Costituzione, pensa e ritiene che le Istituzioni siano cosa loro. *(Applausi)*. Io le avrei chiesto la parola

comprendere come mai l'AIFA, che è un altro pezzo delle nostre Istituzioni, è diventata una sorta di società di consulenza per conto

perché abbiamo chiesto al ministro Schillaci di venire qui, magari con il ministro Nordio, così li prendiamo insieme uno dietro l'altro. Stanno utilizzando pezzi dello Stato per fare per fare pressione e *lobby* attraverso gruppi economici. Lo dico, signora Presidente, perché non consentiamo più

di sapere quando verrà qui il ministro Nordio, esattamente come ha chiesto il Gruppo Partito Democratico a Montecitorio. Abbiamo già depositato un'interrogazione urgente su questa vicenda gravissima, gravissima, che sicuramente sarà oggetto di attenzione dell'autorità giudiziaria, perché una cosa del genere non si è mai vista. Le chiediamo quando verrà qui il ministro Schillaci. Siccome l'unica cosa certa, accanto a questa riforma sgangherata, è che state privatizzando le Istituzioni della Repubblica, fermatevi. Se non vi fermate, lo faremo noi, in ogni caso, con gli strumenti della democrazia garantiti dalla Costituzione che volete calpestare. Senatore Boccia, abbiamo già preso nota di tutti gli interventi e anche della richiesta, che riferiremo, come avevo già detto in precedenza, al presidente La Russa, il quale riferirà, anche perché io non sono in grado di dirle immediatamente l'agenda del ministro Nordio.

intanto chiederei al presidente Zaffini, tramite lei, se può tornare dalla sua parte e consentirmi di parlare. *(Commenti).* Sì, per esempio, direi che è un principio di educazione. Chiedo per esempio, piuttosto che fare il tifo da stadio sotto la curva avversaria, tanto per toccare un tema. Poco fa abbiamo assistito a qualcosa che, se questa riforma se questa riforma dovesse andare in porto, non vedremo più. Abbiamo assistito ad un intervento serio del presidente Pera (che vorremmo ascoltare più spesso, ma che quando parla ascoltiamo comunque volentieri), il quale ha fatto una richiesta molto semplice:

una possibilità di chiarire meglio - ha detto il presidente Pera - quella che può essere la volontà del legislatore.

che quello a cui abbiamo assistito non lo potremo più vedere se questa riforma dovesse andare in porto, per il semplice motivo che un parlamentare non si sognerebbe mai più di andare contro la propria maggioranza, perché sa benissimo di essere in balia del Presidente del Consiglio e di non poter esprimere liberamente la propria opinione. Questo perché quella

quest'Aula. *(Applausi)*. Voi volete impedire qualsiasi formula e modello di rapporto tra il potere legislativo e il potere esecutivo, volete eliminare qualsiasi forma di autonomia. Soprattutto c'è un problema e lo dico, tramite lei, alla ministra Alberti Casellati, che quando avrà finito di parlare col ministro Urso magari ascolterà.

quello che volevo dire alla ministra Casellati è che la cosa che a noi preoccupa, oltre a tutto il testo così come è stato scritto, è che dalle risposte che la presidente Casellati ci dà sembra che la stessa ministra Casellati non abbia ben chiaro che cosa c'è scritto in questa riforma, perché dà delle risposte che non sono attinenti nel merito. Qui tutti i colleghi

È importante perché purtroppo l'esito dei nostri interventi non ha una buona fortuna, ma non ci stancheremo di cercare di capire se questa maggioranza - che con l'atteggiamento che ha avuto fino adesso, purtroppo la risposta se la dà da sola - abbia o no intenzione di entrare nel merito di una riforma costituzionale che viene trattata qui come se fosse una specie di scherzo. L'atteggiamento dell'Assemblea non ha *gravitas*, non c'è serietà, non c'è forma e badate bene, la forma è sostanza. Sembra che stiamo facendo un dibattito al circolo degli amici *(Applausi)*, quando qui siamo in Senato e stiamo affrontando una delle riforme a mio parere più sconclusionate presentate nell'arco di questi ultimi trent'anni sull'assetto costituzionale e istituzionale italiano e ne abbiamo viste tante in Parlamento. *(Applausi).* Mi dispiace dirlo perché mi aspettavo, una volta che è stata presentata una norma come questa, che ci fosse la volontà di entrare nel merito almeno di almeno di quegli aspetti così platealmente fuori dagli assetti delle democrazie liberali e continuiamo a dire questo. Questa riforma costituzionale creerà un Parlamento e un rapporto tra il Parlamento e l'Esecutivo senza contrappesi, senza *check and balance*, che sono presenti presenti in tutte le democrazie liberali, siano esse presidenziali, semipresidenziali, cancellierato alla tedesca o monarchie costituzionali e parlamentari come in Inghilterra. un *unicum*. Il premierato di cui voi vi state riempiendo la bocca sarà ricordato con vergogna da questo Paese. *(Commenti).* State scrivendo la storia, scrivendo voi con queste giornate, con questa sufficienza, con questa supponenza, con questa arroganza, ma gli italiani a un certo punto se ne accorgeranno e vedremo che cosa faranno.

ha spiegato, in termini teorici, e io vorrei provare a farlo in termini pratici e sintetici. Cosa accade? Con l'approvazione dell'articolo 6, che modifica l'articolo 57 della Costituzione, si va ad istituire il premio di maggioranza in Costituzione, garantendo che la coalizione che sostiene la candidatura del Presidente del Consiglio abbia la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento e che quindi, potenzialmente, possa approvare tutto ciò che passa al suo vaglio. Passiamo all'analisi dell'articolo 7, ora in trattazione, che va a modificare l'articolo 94 della Costituzione, aggiungendo dei commi. cosa accade se il Parlamento approva una mozione di sfiducia al *Premier*? Il Presidente della Repubblica ha l'obbligo di sciogliere le Camere. Quindi, se il Parlamento, in particolare la maggioranza (quindi, (quindi, il vostro lato del Parlamento), approva la mozione di sfiducia, praticamente si sta suicidando. Si va tutti a casa, accadrà il suicidio di massa. La seconda ipotesi: se il *Premier* si dimette, può proporre lo scioglimento delle Camere. Di nuovo, il *Premier* si dimette e porta con sé tutti quanti. Quindi, questo è un suicidio di massa o un suicidio insieme ad un omicidio. Terza ipotesi: se il *Premier* si dimette e non scioglie le Camere, il Presidente della Repubblica può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente dimissionario. In questo caso mi sorge il dubbio: ma che maggioranza creerà? Forse sceglierà anche tra parlamentari eletti non nelle liste che hanno sostenuto la sua candidatura oppure un altro parlamentare eletto in collegamento col *Premier*. Qui cosa succede? Il *Premier* ha il diritto di sopravvivere ai parlamentari della coalizione che ne hanno sostenuto l'elezione. Quindi, pur di non morire, il *Premier* il *Premier* uccide la maggioranza che lo ha sostenuto. Quarta ipotesi: se il *Premier* muore, ma questa volta fisicamente, decade o ha un impedimento permanente, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo ad altro parlamentare eletto in collegamento col *Premier*. Qui, invece, il *Premier* fa testamento e fa sopravvivere a se stesso la maggioranza che lo aveva sostenuto. In estrema sintesi, i parlamentari di maggioranza saranno la *longa manus* del *Premier* in Parlamento, a pena della propria sopravvivenza. Quindi, sono di fatto espressione del potere esecutivo

per riguardo a un ex Presidente come il senatore Pera ed anche perché noi, fino all'ultimo, non ci rassegneremo a non entrare al merito delle questioni, io ritengo si debba provare a capire le ragioni per cui il Governo e il relatore darebbero parere negativo a questo emendamento.

molte perplessità sul merito anche dell'emendamento del presidente Pera, ma il problema, prima di pronunciarsi, è capire qual è il significato.

dimissione volontaria e bocciatura di una questione di fiducia. In questa equiparazione ci sta equiparazione ci sta il voler distinguere, come peraltro fa il testo del Governo, l'ipotesi in cui la fiducia venga meno a seguito di una mozione...

Distinguere il caso in cui il rapporto di fiducia venga meno a seguito di una mozione del Parlamento dal caso in cui il rapporto di fiducia venga meno venga meno a seguito di una bocciatura da parte del Parlamento di una questione di fiducia è sempre un atto del Parlamento che interrompe il rapporto fiduciario. Come si può immaginare una diversa disciplina a seconda che ci sia la mozione o ci sia la bocciatura di una questione di fiducia?

o meglio di dimettersi ma di chiedere al Presidente della Repubblica un nuovo incarico. Come si può distinguere queste due ipotesi? C'è sempre un'interruzione del rapporto di fiducia da parte...

normale incidente per cui c'è qualche numero in meno, come può succedere nella vita normale di un Governo, per cui magari si va sotto su un decreto perché quel giorno ci sono delle assenze oppure dei senatori in missione. Stiamo parlando di due fattispecie molto simili, quelle che venivano richiamate

due sbocchi diversi (perché in un caso c'è lo scioglimento delle Camere e nell'altro caso invece c'è la possibilità della concessione di un nuovo incarico) sembra davvero una cosa del tutto incomprensibile. Ancora una volta, anche su questo punto, se ci fosse da parte del Governo perlomeno un elemento di precisazione su una cosa che peraltro tantissimi costituzionalisti che abbiamo audito nel corso dei mesi scorsi hanno obiettato un elemento perlomeno di poca certezza o comunque di straniamento rispetto alla questione, penso che sarebbe davvero opportuno. non ci sia, da parte del Governo e della maggioranza, una precisazione mi sembra abbastanza singolare. Torno pertanto a chiedere alla Ministra o al relatore se fossero così gentili da spiegare come si distinguono queste due fattispecie e perché in un caso c'è un *iter* previsto e in un altro caso ce n'è un altro. Davvero viene il dubbio che questa cosa sia frutto di una sintesi fatta male. non ci giriamo intorno: noi lo sappiamo dall'inizio che su questo punto specifico c'è un dissenso tra le forze di maggioranza perché Fratelli d'Italia era favorevole al *simul simul*, come sappiamo, la Lega no e io penso ho finito davvero - che il frutto pasticciato di questo aspetto che è stato richiamato dal senatore Giorgis e che io ho voluto riprendere, abbia probabilmente a che fare con questo. Come si vede, quando si fanno le mediazioni male e si cerca di conciliare punti di vista che non necessariamente sono conciliabili, poi si finisce col mettere in campo una norma che è totalmente discutibile e che, al di là della polemica politica che si può fare in quest'Aula, come è normale che sia, obiettivamente mette in evidenza elementi totalmente incomprensibili.

dopo l'intervento della ministra Alberti Casellati mi assale veramente un dubbio e credo molto a questo confronto; nonostante sia così mancato,

il potere passa - ad oggi, a Costituzione vigente - nelle mani del Presidente della Repubblica che valuta il quadro e indirizza un po' la situazione. Oggi è così. Di fronte a questo articolo, per come lo votiamo - i nostri emendamenti vanno esattamente in questa direzione - ci piaccia oppure no, è proprio evidente che la scelta sta unicamente nelle mani del Presidente del Consiglio, che da questo punto di vista tiene sotto ricatto il Parlamento, perché sarà solo il Presidente del Consiglio che deciderà con le dimissioni che consegna nelle mani del Presidente del Repubblica, che non avrà alcuna scelta qualora si dimettesse. Qualora si dimettesse, il Presidente della Repubblica dovrà sciogliere le Camere. *(Applausi)*. Allora è vero che cambiano o non cambiano i poteri del Presidente della Repubblica? Me lo chiedo solo per chiarezza tra noi e perché non sia veramente un dialogo tra sordi. È così chiaro che cambia

noi abbiamo ascoltato le argomentazioni del Presidente di Commissione e della Ministra sui pareri all'articolo 7 ben più lunghe, ma comunque a finire oggetto delle caricature del Governo è stata questa volta la figura del Capo dello Stato, che invece non dovrebbe essere tirata in mezzo così come è stato fatto. Si continua a dire che i suoi poteri di garanzia non vengono toccati, invece vengono completamente svuotati, ed è bene sapere che le emergenze istituzionali non si possono abolire per decreto. Volevate abolire per decreto la scorsa settimana le liste d'attesa; non si poteva fare; non si possono abolire nemmeno le emergenze politiche. Possono capitare, anche con questa riforma costituzionale, e, se capitano, è bene che il Capo dello Stato possa prestare la sua autorevolezza per la ricerca di una soluzione. Nel nostro ordinamento il Capo dello Stato aiuta a trovare soluzioni e non può imporre niente. Voi, con questa riforma, gli togliete qualsiasi possibilità di agire nelle emergenze per favorire delle... *(Il

Signora Presidente, provo a proseguire da dove è stato interrotto il presidente Parrini. Noi abbiamo deciso la Repubblica - torno su una cosa che ho già detto in quest'Aula - dopo aver fatto un *referendum* che sceglieva tra la Repubblica e la monarchia. il Paese ha scelto la Repubblica esattamente immaginando di non ricostruire una situazione in cui ci fosse un potere unico nelle mani, in quel caso, di una dinastia o di una singola persona. Qui ci ritroviamo esattamente nella situazione che stiamo ricostruendo un qualcosa che nega il presupposto della nostra Costituzione, cioè che il potere è nella Repubblica parlamentare, per dire che invece c'è una persona che può determinare quali sono le sorti. A me continua a stupire il fatto che non vi rendiate conto che le prime vittime di questo processo sono gli eletti e i rappresentanti nel Senato e nella...

La materia effettivamente è abbastanza complessa. Vi dico che, se io fossi l'avvocato dei parlamentari di maggioranza, sarei preoccupata, nel senso che vi direi di fare attenzione, perché state sottoscrivendo un contratto che non vi vede parti favorite, anzi vi vede parti calpestate. Mi chiedo se voi abbiate le idee chiare e se stiate sottoscrivendo questo patto consapevolmente. E mi stupirebbe.

Signora Presidente, mi pare che sull'argomento siano evidenti due cose fondamentali. La prima è che la nostra proposta alternativa era chiarissima: la sfiducia costruttiva, che voi non avete preso in considerazione.

Facciamola una riflessione, leggendo semplicemente il testo, perché lì vediamo come il Presidente della Repubblica diventa il servo sciocco, cioè quello che, tutto sommato, è un esecutore di ordini. In caso di revoca della fiducia il Presidente della Repubblica scioglie scioglie e non ha nessun tipo di intervento. E ci siamo. Ma anche in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, se e solo se il Presidente del Consiglio può proporre entro sette giorni lo scioglimento delle Camere. E il Presidente della Repubblica che fa? Il Presidente del Consiglio può valutare, può fare tutte le analisi, esprimere tutte le considerazioni del caso e il Presidente della Repubblica cosa fa? Il Presidente della Repubblica dispone. Il Presidente della Repubblica dispone. State facendo diventare il Presidente della Repubblica uno che esegue semplicemente gli ordini *(Applausi)* e questo non è bello. Questo vi autorizza sicuramente a dire che questa è la madre di tutte le riforme, però siete però siete pregati di non dire due cose. In primo luogo non trovate termini di paragone con altri ordinamenti costituzionali stranieri perché non ne troverete uno pari alla schifezza che avete scritto! *(Applausi)*. Non ne troverete uno.

Francia; questa roba qui non la troverete da nessuna parte. E fatevela una domanda. *(Commenti)*. In secondo luogo non vi azzardate a dire che non state toccando i poteri del Presidente della Repubblica perché il Presidente della Repubblica tra pochi minuti diventerà il servo sciocco del vostro *Premier*!

perché mi vedo costretto, e cerco di farlo con la massima pacatezza e in modo niente affatto provocatorio, a chiedere che la Presidente del Consiglio intervenga qui in Senato,

qual è il rapporto che questo Governo e questa maggioranza intendono costruire con alcune delle pagine più vergognose della nostra storia. Spiego perché faccio questa richiesta.

sull'autonomia differenziata.

era avvenuto un fatto gravissimo come l'esibizione del simbolo della Decima Mas in Aula. Pochi giorni fa noi abbiamo fatto un'interrogazione alla quale non è stata data alcuna risposta. Lei avrà letto che il Governo ha autorizzato l'emissione di un francobollo, dedicato a onorare la memoria di Italo Foschi.

mi bastano, altrimenti non mi bastano. Concludo dicendo che è stato dedicato un francobollo a Italo Foschi, cioè a uno dei peggiori e più violenti esponenti dello squadrismo romano. Siamo finiti sul «Financial Times»; il ministro Urso, in preda all'imbarazzo, non ha partecipato…

Aula)*. Senatore Parrini, io non ho paura della verità, ma lei si è preso tre minuti e non sono ancora riuscita a capire qual è la richiesta sull'ordine dei lavori. lavori. Facciamo così: io le do un minuto, se lei ce la fa va bene, altrimenti passo al voto. Chiedo alla maggioranza, per cortesia, di fare silenzio in questo minuto in cui finalmente capiremo qual è la richiesta sull'ordine fuori, perché io ancora non l'ho capita. volevo finire di spiegare che il ministro Urso, in preda a grave imbarazzo dopo l'uscita dell'articolo sul «Financial Times», ha deciso di non partecipare alla cerimonia di celebrazione di questo francobollo (con una decisione saggia che io apprezzo, perché sapersi vergognare è importante), ma non ha ancora ordinato l'incenerimento di quella emissione filatelica. Quel francobollo dedicato a uno squadrista deve essere incenerito e quindi la Presidente del Consiglio… *(Il microfono si disattiva automaticamente.).*

a una riflessione. Io non so se ci si sta rendendo conto del clima che accompagna questa riforma e anche di parole molto bugiarde che si sono sentite in quest'Aula, le più gravi delle quali sono arrivate dal Governo. Continuare a ripetere agli italiani che il ruolo del Presidente della Repubblica non viene toccato è una palese bugia, ma io credo che noi dobbiamo, prima di procedere, interrogarci interrogarci davvero e provare a ricordarci quanto è valso in questi anni il ruolo e il peso che il Presidente della Repubblica ha messo nella soluzione e nella ricerca di soluzioni per questo Paese, non per la maggioranza.

Vorrei ricordare che il Governo ha giurato sulla Costituzione italiana antifascista, ma questa riforma scellerata, insieme a tutte le altre che che abbiamo visto e che si ventilano (tipo l'attacco al potere giudiziario, che dev'essere sottoposto al controllo dell'Esecutivo; l'imbavagliamento del Parlamento, che con questa riforma viene sottoposto al potere esecutivo; la riduzione di tutte le prerogative della figura di garanzia che è il Presidente della Repubblica, sempre ad opera di questa riforma, che smantella tutta la Costituzione nei suoi pesi, contrappesi e bilanciamenti), mi sembra denoti un chiaro atteggiamento, nella pratica, fascista.

Siccome pochi minuti fa, nel suo intervento, ci ha accusati di essere strumentalizzati dai terroristi e dai mafiosi, voglio chiedere formalmente al presidente Balboni, che in quest'Aula dovrebbe essere anche il Presidente di una Commissione e dunque garante del rapporto con le opposizioni, di chiedere formalmente scusa a quest'Assemblea e soprattutto di chiedere a quest'Assemblea il ritiro di una espressione inaccettabile. Le voglio ricordare, Presidente, che noi abbiamo sempre fatto della lotta alla mafia e della legalità le nostre radici e i nostri princìpi. *(Applausi)*. Non vorrei che stessimo interpretando questa modifica...

di intervenire in maniera ufficiale affinché siano smentite le accuse che ci sono state rivolte. Noi non abbiamo niente a che fare con queste aggressioni.

gerarchi e *kapò* in quest'Aula che usano gli strumenti dell'illegalità per accusare le opposizioni.

ciò non riguarda i nostri lavori. Siamo in Senato e non riguarda questi lavori.

In un gesto dimostrativo, un deputato del MoVimento 5 Stelle ha semplicemente portato

portato via in carrozzella. Questa è una violenza squadrista inaccettabile nelle Aule più sacre della democrazia. È questo è il vostro modo di comportarvi a tutti i livelli? È vergognoso! Questa violenza va arrestata e quest'arroganza va fermata. Riflettete e vergognatevi!

State abdicando ai vostri diritti di parlamentari, ma questo poco mi interesserebbe, se non fosse che la vostra abdicazione poi coinvolge tutto il resto dei parlamentari. Non è una cosa accettabile. Mi chiedo alla luce di quale obiettivo finale stiate abdicando ai vostri diritti, ai diritti del Parlamento italiano e, in ultima analisi, ai diritti di tutti gli italiani.

Il premieriato vuole che, se c'è una mozione di sfiducia motivata, il Presidente della Repubblica sciolga il Parlamento. Se c'è una dimissione volontaria oppure dimissioni a seguito di mancanza di di fiducia su un provvedimento, il Presidente del Consiglio ha tre possibilità:

finito il quale il Presidente ha sette giorni di tempo per andare dal Presidente della Repubblica ed esperire le tre possibilità. Su questa scansione dei tempi è d'accordo il Governo ed è d'accordo il relatore. La prima fase è quella che ho chiamato parlamentarizzazione della crisi, che già sarebbe un grande risultato rispetto all'esperienza che abbiamo avuto in tutti questi anni dal dopoguerra. La seconda fase, invece, sono le decisioni del Presidente del Consiglio e le comunicazioni al Presidente della Repubblica. La prima fase prevede l'informativa del Presidente del Consiglio. La domanda è: informativa su che cosa? Sulla crisi e sulle ragioni della crisi. È venuta a mancare la maggioranza e il Presidente del Consiglio, per ragioni sue insindacabili, decide di dimettersi. L'informativa, ovviamente, non riguarda le fasi successive (le quali possono essere scioglimento del Parlamento, reincarico oppure passaggio della mano), ma solo le ragioni della crisi. Osservo che nel modo in cui è scritto il testo del Governo, che pure intende rispecchiare questa successione di fasi, esiste margine di ambiguità. Le lingue naturali hanno questi margini sempre. Non sono linguaggi simbolici e quindi hanno questo margine. Sembrerebbe, secondo un'interpretazione magari un po' forzata, che che l'oggetto dell'informativa da parte del Presidente del Consiglio che si dimette sia la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere, ciò che non è, non ha in mente il Governo e non ha in mente il relatore. Allora ho riformulato la norma semplicemente in un italiano diverso, credo un po' più semplice, questa successione delle fasi: l'informativa del Presidente del Consiglio, nel caso di dimissioni, riguarda la natura delle dimissioni e le prospettive della crisi. Tutto qua. Penso che sia un emendamento neanche di sostanza, ma la riformulazione linguistica di un'espressione contenuta nel testo del Governo, che rispecchia lo stesso stato di cose, cioè la successione di fasi a cui ho fatto riferimento. Ecco perché raccomando questo emendamento.

però mi associo naturalmente alle sue argomentazioni e alla richiesta al Governo e al relatore di accogliere questo emendamento perché, appunto, spiega meglio come si dovranno svolgere le fasi successive alla caduta del Governo, alle dimissioni,

che nel corso dell'informativa il *Premier* venga qui e chieda lo scioglimento delle Camere; è così, senatore Pera, e in effetti è vero. è vero. In questo momento abbiamo l'eventualità, a meno che non vogliate porvi rimedio, che effettivamente ci sia un passaggio nelle Camere e nel corso dell'informativa,

che è evidente che, così com'è scritto, l'informativa riguarda il potere di scioglimento e non la parlamentarizzazione della crisi. Mi sembra abbastanza evidente. Quello che chiede il presidente Pera è una questione di buonsenso e non capiamo il motivo per cui il Governo insista con un parere non lo capiamo per la forma, non lo capiamo per il contenuto e non lo capiamo soprattutto perché rileviamo anche una mancanza di rispetto per una persona che è stata Presidente del Senato e che cerca di contribuire al miglioramento di una riforma pasticciata. Ammiriamo lo sforzo del presidente Pera. Mi sa che questa è davvero una missione impossibile.

Signora Presidente, l'emendamento che aveva proposto il presidente Pera è assolutamente di buonsenso. Ho notato che è stato condiviso da sei parlamentari della maggioranza.

Presidente, in questi lunghi giorni di discussione sulla riforma cosiddetta del premierato, ho chiesto

Signor Presidente, voglio ricordare in quest'Aula il senatore Alberto Robol, scomparso a Trento lo scorso 29 maggio. Robol ha cominciato a fare politica da giovanissimo nelle file della Democrazia Cristiana, ricoprendo tutti gli incarichi del movimento giovanile, fino alla segreteria provinciale. Tra i fondatori del Partito Popolare Italiano, ne è stato segretario provinciale. Nel 1998 viene eletto in Consiglio provinciale, incarico che poi lascia una volta proclamato senatore nel 1991. Da quel momento, siederà tra questi banchi per tre legislature, fino al 2001. Per molti anni Robol è stato uno dei protagonisti della tradizione cattolico-democratica del Trentino, che ha declinato attraverso una politica dell'ascolto, della costante apertura al dialogo in proposte mai banali e in visioni sempre lungimiranti. Grande oratore, ha appassionato generazioni di giovani alla politica, anche attraverso il gruppo Don Milani di Trento, in cui si sono formati diversi esponenti politici divenuti poi parlamentari in rappresentanza del Trentino e in vari partiti. Ha certamente contribuito alla trasformazione culturale ed economica del Trentino fin dai primi anni Sessanta nel mito di John Fitzgerald Kennedy, di cui era un grande estimatore, e lo ha saputo fare in anni di profondi cambiamenti che, come sappiamo, impattarono in maniera molto forte sull'esperienza dei cattolici in politica. Robol non subì però passivamente questi cambiamenti. Da uomo cresciuto alla scuola di Aldo Moro, che considerava il suo maestro politico e il riferimento ideale, ne colse il senso e accettò la sfida per rinverdirli nell'idea che era finito sì il partito dei cattolici, finite la funzione e le ragioni storiche del loro ruolo in politica. Chiusa l'esperienza nelle istituzioni, il suo impegno per la comunità è proseguito per ben come reggente della Fondazione Opera Campana dei caduti, dando lustro e prospettiva internazionale a questa importante istituzione di pace del nostro territorio. I tanti messaggi di cordoglio di questi giorni e il ricordo delle persone a lui vicine, degli amici come degli avversari politici, sono la cifra delle sue qualità politiche, umane e culturali. Il Trentino ha perso una figura preziosa, ha perso un uomo di pace e quante ce ne vorrebbero adesso di figure come Alberto Robol, in un tempo nel quale, anche nella nostra Europa, la pace ha smesso di essere il bene supremo. Per questo lo piangiamo e ci stringiamo al dolore dei suoi cari e dei tantissimi che gli hanno voluto bene.